Onorevoli colleghi, come vi è ormai tristemente noto, nel cuore di questa notte una violenta esplosione, provocata dal deragliamento di un treno merci carico di gas, seminato morte e distruzione intorno alla stazione ferroviaria della città di Viareggio. Alcuni edifici sono stati investiti dall'esplosione e dalle fiamme che si sono immediatamente propagate, provocando numerose vittime, il cui numero totale, al momento, supera purtroppo di gran lunga la decina. I Vigili del fuoco e le squadre dei soccorritori, prontamente accorsi anche dalle città vicine e da tutta la Regione, dopo aver lottato tutta la notte contro il fuoco, stanno ora scavando tra le macerie alla ricerca di superstiti. Sono certo di esprimere il sentimento di tutta l'Assemblea nel rivolgere, ancora una volta, un commosso ringraziamento al Corpo dei Vigili del fuoco e agli uomini e alle donne della Protezione civile, delle forze dell'ordine, dei servizi sanitari, nonché a tutti i privati cittadini che, anche in questa dolorosa occasione, si sono volontariamente messi a disposizione delle autorità per collaborare a salvare il maggior numero possibile di vite. Non è certamente questo il momento delle polemiche; sarà però necessario, nei prossimi giorni, accertare con rigore tutte le eventuali responsabilità connesse al verificarsi di questo gravissimo incidente, affinché le istituzioni competenti - già da ora operanti - siano in grado di offrire una risposta esauriente e soddisfacente su quanto accaduto. Lo dobbiamo non soltanto alle tante famiglie così duramente colpite dal lutto e dalla devastazione, ma anche a tutto il personale dei trasporti ferroviari, che chiede di essere rassicurato circa le condizioni di sicurezza nelle quali quotidianamente si svolge il suo delicato e importantissimo lavoro. Il Governo si è prontamente dichiarato disposto a riferire nell'Aula del Senato fin dalla giornata di domani, non appena in possesso di tutti gli elementi necessari per una prima, informata risposta. In segno di cordoglio per le vite spezzate da questa immane tragedia, tra le quali si contano purtroppo diversi bambini, e di vicinanza della nostra Istituzione alle sofferenze della popolazione di Viareggio, sentimenti accompagnati naturalmente dal sincero augurio di un pronto ristabilimento per tutti i feriti, invito l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento.

Come sempre, Vigili del fuoco e Protezione civile sono prontamente intervenuti contenendo i danni e limitando l'entità di un bilancio di per sé tragico. A loro rivolgo un incoraggiamento, un apprezzamento e un sostegno non rituale. Questo nostro Paese subisce con fatale regolarità l'accanirsi di drammatici e tragici eventi, spesso imprevedibili, ma che a volte nascondono colpe e trascuratezze inaccettabili per un Paese avanzato.

Questi sono momenti da dedicare ad alleviare le sofferenze di chi è stato colpito e a ripristinare, nel più breve tempo possibile e in tutta sicurezza, condizioni di vita, di lavoro e di trasporto nella città di Viareggio. Più avanti dovremmo tutti porci interrogativi seri e, soprattutto, fornire risposte pertinenti e all'altezza dei tempi sul trasporto in Italia e sui livelli di sicurezza del trasporto pubblico. Se da un lato è giusto sottolineare i risultati raggiunti in alcuni comparti di punta del nostro sistema ferroviario, non è tuttavia tollerabile che il complesso del servizio ferroviario venga trascurato e lasciato deperire, sia in termini di qualità che di sicurezza. Lasciatelo dire ad un uomo del Sud che vive sulla propria pelle l'arretratezza mostruosa dell'apparato infrastrutturale ferroviario del nostro Mezzogiorno e delle Isole. a poche settimane or sono un altro incidente ferroviario, dovuto sempre alla rottura di un asse di un carrello, che ha bloccato per più di 24 ore la linea Bologna-Firenze, ossia il cuore del trasporto ferroviario nazionale. Certo, un incidente non paragonabile neanche lontanamente a quello di Viareggio per l'entità del disastro, anche in termini di vite umane, e la pericolosità dell'evento. Si tratta, comunque, di un segnale che ci dice che il nostro sistema dei trasporti ferroviari, certamente complesso e articolato, è probabilmente vecchio ed obsoleto

al materiale esplosivo e altamente pericoloso che attraversa, con una concentrazione così elevata, zone così intensamente abitate sia lungo la linea adriatica, che lungo la dorsale tirrenica. Si parla di 14 vagoni di GPL contenuti in un solo convoglio che subisce un deragliamento, presumibilmente per la rottura di un carrello, in pieno centro di una importante città rivierasca. Sono poi necessari interventi ordinari per garantire la sicurezza e la regolarità del trasporto pubblico. I cittadini hanno il diritto di prendere il treno sicuri che il servizio sia all'altezza di un Paese civile valere per tutti i cittadini, sia per chi si sposta per lavoro o per vacanze, ma a maggior ragione per i lavoratori pendolari che il treno sono costretti a prenderlo sempre, tutti i giorni. Le risorse messe a disposizione delle Ferrovie da parte dello Stato rappresentano una fetta molto consistente delle risorse pubbliche che annualmente vengono spese per migliorare e garantire servizi ad un grado accettabile di civiltà. Si può discutere se le risorse messe a disposizione siano adeguatamente sufficienti, ma è tuttavia probabile che vengano spese male privilegiando settori da portare come fiore all'occhiello (ad esempio, l'alta velocità) e trascurando settori altrettanto importanti, come il trasporto locale e la sicurezza nel trasporto di merci, specie se pericolose, settori che sono andati sempre più deperendo in termini di qualità, di sicurezza e di manutenzione ordinaria. A fronte di questi pochi e affrettati spunti, che serviranno poi per l'avvio di una più approfondita discussione sui temi del trasporto e della sicurezza, ora il momento di rivolgere il nostro pensiero commosso a chi soffre, a chi ha perso la vita e i propri beni in questa tragedia, augurandoci di giungere al più presto a chiarire in modo certo e giusto le cause di quanto è avvenuto. Signor Presidente, anche noi ci associamo alle sue parole di cordoglio nei confronti delle famiglie delle vittime e dei feriti della tragedia di Viareggio tragedia di Viareggio ed esterniamo la nostra vicinanza alla città di Viareggio, che ha subito questa tragedia immane e profondamente lacerante.

materiale altamente infiammabile e che si trovava nel centro della città di Viareggio. *(Brusìo)*. PRESIDENTE. Colleghi, posso chiedervi una maggiore attenzione su questo tema e, in genere, in Aula?

e quant'altro. È necessario far luce su questa vicenda - come lei giustamente ha detto, e noi siamo d'accordo - e avviare un'inchiesta amministrativa impietosa, per accertare fino in fondo se e in che misura vi siano responsabilità in ordine a episodi di questa natura.

non solo e non tanto a quella che si sta ammodernando con il sistema dell'Alta velocità e dell'Alta capacità, quanto a quella rete ferroviaria che rappresenta la spina dorsale dei trasporti del nostro Paese e che viceversa è abbandonata a se stessa.

che la rete di trasporto locale attraversa tante città, tanti centri cittadini, dobbiamo capire qual è la politica che Ferrovie dello Stato intende o ha inteso applicare per garantire la sicurezza del trasporto, almeno

DE TONI *(IdV)*. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, in una notte da poco estiva, in una solare e gioiosa cittadina della Versilia, Viareggio, irrompono la morte, il dolore, la sofferenza. Perché? È davvero colpa dell'imprevedibile o è forse responsabilità dell'incuria, della disattenzione, del pressappochismo? Questa notte è successa una tragedia immane, che ha colpito 13 vittime innocenti. Questo, almeno finora, è il numero dei morti accertato, cui si aggiungono decine e decine di feriti; tra le vittime vi sono tre bambini. Appena un paio d'ore fa, abbiamo saputo che è stata trovata un'altra bambina, una piccola di quattro anni, e purtroppo il bilancio sembra destinato a crescere, visto che numerose persone risultano ancora disperse. Ci auguriamo che non sia così. Come in ogni tragedia, però, anche in circostanze terribili come questa, dobbiamo cogliere i pochi segni di speranza: così, abbiamo appreso che questa notte, dalle macerie di una palazzina crollata in conseguenza dello scoppio, sono state estratte ancora vive altre persone, altri bambini. Un piccino di tre anni è stato estratto vivo dalle macerie poco fa. Noi dell'Italia dei Valori, prima di tutto, vogliamo stringerci attorno alle famiglie che hanno perso i propri cari e a quelle che sono in apprensione per i propri parenti in ospedale, alcuni dei quali versano in condizioni gravissime. A questi facciamo i nostri auguri per una guarigione il più possibile rapida. Ma lo dico ancora: una tragedia come questa, ogni tragedia, può essere evitata, cari colleghi del Senato La magistratura, che ha cominciato immediatamente le proprie indagini, ci dirà se anche questa volta esistono particolari responsabilità da addebitare a persone o ad imprese, vi sono state colpe nella manutenzione delle carrozze, come starebbe emergendo - il condizionale è d'obbligo - dalle prime confuse notizie. Seguiamo con grande rispetto il lavoro degli inquirenti e, come nostro costume, non interferiremo. Oggi è il giorno del dolore e del lutto, non è il caso di lanciare accuse, che pure avremmo voglia di lanciare, perché di fronte alla rabbia per una tragedia di queste dimensioni vengono in mente tutte le volte in cui, Cassandre inascoltate, abbiamo denunciato i tagli di bilancio, a nostro parere inopportuni proprio perché andavano ad incidere, tra le altre cose, sulla sicurezza delle nostre ferrovie, su cui ogni giorno viaggiano milioni di persone. Non osiamo immaginare le conseguenze di questo incidente se lo scoppio fosse avvenuto in pieno giorno! Ma oggi, dicevo, è il giorno del lutto. Dunque, le polemiche le lasciamo ad altri: badate bene, neanche di fronte a tragedie come questa perde il pessimo vizio di criticare la parte politica avversa, come ha fatto questa mattina il presidente del Consiglio Berlusconi a Napoli. L'Italia dei Valori sa che ci sono giorni per riflettere e giorni per denunciare. Oggi abbiamo solo voglia di riflettere su quello che poteva essere e non è stato, su tante persone che soffrono e su cosa possiamo fare perché tragedie di questa portata non accadano mai più. Signor Presidente, colleghi, il disastro di oggi a Viareggio è stato preceduto nel mese di giugno da altri due incidenti avvenuti sempre in Toscana, fortunatamente senza vittime. Il bilancio di quest'ultimo incidente è invece, purtroppo, pesante: finora 14 morti e molti altri feriti gravissimi. In attesa di verificare le cause precise di questa orribile tragedia, verifica affidata alla magistratura e alla Commissione d'inchiesta che il ministro Matteoli intende costituire, alcuni interrogativi cominciano ad affiorare circa i controlli sui mezzi che trasportano materiali pericolosi e i componenti dei medesimi, prodotti spesso da soggetti diversi. Si discute dell'opportunità di aggiornare alcune norme di sicurezza anche a livello europeo, basandole sul principio dei chilometri percorsi più che sul tempo trascorso tra i successivi controlli. La liberalizzazione nel settore dei trasporti, se può favorire i mercati di fronte alla maggiore competitività delle tariffe, non deve e non può andare a discapito della sicurezza e dei controlli stessi. Oggi, comunque, non è certo il giorno delle polemiche né quello di invocare colpe a carico di qualcuno, ma neanche di rinunciare a programmi di ammodernamento dell'Alta velocità. Certo è che la dinamica dell'incidente lascia attoniti ci si chiede se forse non si debbano fare maggiori investimenti in sicurezza ad ogni livello nel nostro Paese, nelle costruzioni, nei trasporti, sui luoghi di lavoro. Una delle emergenze nazionali è certamente la sicurezza.

*(PD)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, 17 morti, di cui tre bambini, decine di feriti tra cui 15 gravissimi, 1.000 abitanti evacuati: questo il bilancio, purtroppo ancora provvisorio, della sciagura di Viareggio. Si tratta di un bilancio tragico, di uno dei peggiori incidenti ferroviari del nostro Paese. Alle vittime va la solidarietà e l'affetto dei senatori del Partito Democratico; ai soccorritori e ai Vigili del fuoco tutta la nostra riconoscenza per l'applicazione e la professionalità con cui sono intervenuti. È nostro dovere da subito riflettere sulla tragedia di Viareggio, capire che cosa è avvenuto; dobbiamo subito dissipare un dubbio, che è emerso anche negli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Il dubbio è che le Ferrovie investano in tecnologie innovative sull'Alta velocità, lasciando a livello di Terzo mondo i servizi per i pendolari ed il trasporto per le merci. Questo il dubbio che dobbiamo dissipare al più presto. Infatti, se l'incidente appena avvenuto è il peggiore della storia recente delle Ferrovie, non è purtroppo un caso isolato. In questi mesi si sono ripetuti altri casi allarmanti, per fortuna senza conseguenze tragiche; casi che ripropongono con forza gli interrogativi in ordine agli standard di sicurezza delle nostre Ferrovie; standard oggetto più volte di interpellanze del Partito Democratico, cui si è sempre risposto negando l'esistenza del problema. Secondo una prima ricostruzione, la causa andrebbe ricercata nel cedimento strutturale di un carrello. dello Stato Mauro Moretti ha detto che si è spezzato l'asse. Secondo la denuncia dei delegati dell'assemblea nazionale dei ferrovieri si tratta di un incidente tipico. Questo aggettivo è particolarmente preoccupante nel senso che esso si è ripetuto innumerevoli volte; da ultimo, nei giorni scorsi, sempre in Toscana, a Pisa-San Rossore ed a Prato. Di fronte a queste prime spiegazioni il nostro allarme aumenta perché sono ricostruzioni che pongono in dubbio l'efficienza dei sistemi e dei controlli di sicurezza. Ringrazio il presidente Schifani dell'invito al Governo a riferire, già domani, su questi fatti, e colgo l'occasione per proporre alcuni quesiti quali sono gli standard di sicurezza dei vagoni che trasportano merci pericolose e, come nel caso in questione, liquidi infiammabili. Secondo: di chi è la responsabilità di verificare l'idoneità all'uso dei vagoni merci. se corrisponde al vero quel che ha affermato la direzione delle Ferrovie che la revisione del carro incidentato prevista dalle normative europee era stata svolta regolarmente. quali sono le responsabilità della società austriaca GATX, proprietaria del vagone incidentato, che oggi ha già cominciato a fare lo scaricabarile sulle proprie responsabilità. Quinto: cosa fa di norma l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria per prevenire incidenti di questo genere, se è vero che si ripetono di frequente. Credo che un'informativa da parte del presidente dell'Agenzia sia indispensabile. chiediamo che provvedimenti intenda adottare il Governo per prevenire in futuro incidenti simili. Chiediamo quindi che il Governo venga in Aula al più presto per rispondere a tali quesiti e per dare una chiara illustrazione delle cause di questa immane tragedia. In un paese civile, ha detto Emma Marcegaglia, queste cose non debbono succedere; lo ripetiamo anche noi: non debbono e non possono succedere. Signor Presidente, anche da parte nostra desideriamo esprimere il più vivo cordoglio per le vittime di questo drammatico incidente e la nostra convinta solidarietà

Le commissioni d'inchiesta che il Governo ha già nominato ritengo avranno modo e tempo per chiarire tutto ciò che c'è da chiarire in questo incidente, che sicuramente, fin d'ora, potremmo definire raro nella sua meccanica. Raro perché, secondo quanto acquisito, il treno procedeva ad una velocità normale, a meno di 90 chilometri all'ora; raro perché nessun lavoratore sui binari è rimasto coinvolto, i macchinisti sono illesi le verifiche fatte dai tecnici delle Ferrovie (secondo dichiarazioni dei vertici delle Ferrovie) sono risultate, alla partenza, assolutamente regolari. La locomotiva del convoglio è rimasta in piedi, i carri di coda sono rimasti intatti sui binari, il sistema frenante non sembra sia dovuto scattare perché non ve ne era bisogno

Sembra, così si dice, ed questa l'ipotesi che sta prendendo piede, che ci sia stato un cedimento strutturale di uno dei 14 carri, in particolare il primo, dopo la locomotiva. A chi in questo momento sottolinea con forza la necessità di andare a verificare se le manutenzioni vengono effettuate regolarmente e puntualmente e se gli investimenti in tecnologia della sicurezza in questi anni sono stati effettuati in modo adeguato, voglio ricordare che la nostra Commissione si è occupata tante volte di tali problemi. È anche per questo motivo, per via di un'azione che il Parlamento ha svolto, che possiamo ricordare a tutti che che soltanto negli ultimi cinque anni le Ferrovie hanno investito non meno di 4,5 miliardi di euro in tecnologia della sicurezza. Vogliamo inoltre ricordare (anche se, in considerazione

la dinamica dell'incidente sia chiarita nel modo più puntuale e veloce, così come eventuali responsabilità. In questo senso, anche noi esprimiamo apprezzamento per il fatto che il Governo si è dichiarato disponibile a venire in Aula per riferire entro la giornata di domani.

di condoglianze e solidarietà verso tutte le famiglie colpite da questo tragico evento. Consentitemi di non aggiungere altro perché il ministro Matteoli - che, come sapete, era all'estero - si è attivato immediatamente per costituire una commissione d'inchiesta, è rientrato immediatamente in Italia, si è già recato sul posto e si è impegnato a riferire,

Lo faccio in un momento di particolare amarezza personale, dichiarando la grande soddisfazione che ho nel condurre a termine un impegno cominciato lo scorso anno,

continuare a comandare dall'interno delle carceri sui territori in cui le mafie svolgono la loro drammatica attività, la quale rappresenta un cancro della società nella quale viviamo. Inoltre, abbiamo rafforzato i poteri di accesso e di accertamento dei prefetti in materia di appalti; anche per la trasparenza ed una maggiore penetrazione nelle amministrazioni locali, coinvolgendo nei provvedimenti non soltanto il personale degli eletti, ma anche i dirigenti dei Comuni che spesso sono quelli che restano, essendo radicati nell'*habitat* mafioso, quando le amministrazioni vengono sciolte. Credo che, unendo lo sforzo di questo provvedimento con quello compiuto con il decreto-legge approvato lo scorso anno, finalmente raggiungeremo un risultato consapevolmente importante nella lotta alla criminalità organizzata. all'inizio del mio intervento - in un momento di particolare amarezza personale: ho voluto tuttavia illustrare il frutto di un lavoro iniziato nei mesi scorsi, nella convinzione che sia nostro compito liberare il Paese dal cancro della mafia anche quando ci si imbatte nella violenza di chi, anziché sparare, cerca con l'infamia e la calunnia di spegnere la voce e l'impegno di chi lavora per restituire allo Stato i beni dei mafiosi, e soprattutto - lo sottolineo - dei loro eredi, e per assicurare per sempre al carcere duro impenetrabile boss che pensano di poter continuare a comandare impunemente le loro organizzazioni. e forse ho violato il Regolamento, signor Presidente, perché ho parlato di provvedimenti che l'altro ramo del Parlamento non aveva modificato e lo stesso Governo non aveva ritenuto di modificare rispetto alla primitiva approvazione da parte del Senato.

abbiamo ritenuto opportuno che il senatore Vizzini prendesse la parola per primo, in quanto l'articolo 2 del disegno di legge concerne nel suo insieme disposizioni in materia di contrasto alla criminalità organizzata

Con il senatore Vizzini abbiamo portato avanti, con il supporto e il contributo dell'opposizione in sede di prima lettura, un'importante iniziativa che andava a completare il pacchetto sicurezza approvato dal Governo in Consiglio dei ministri. Si trattava di dare una risposta immediata alle attese del popolo italiano, il quale giustamente aveva posto la questione sicurezza come prioritaria rispetto a tutte le altre questioni, sia pure importanti, che pesavano sui cittadini e sul popolo del nostro Paese. Il Governo e il Parlamento hanno dato risposte rapide, efficaci e condivise dall'opinione pubblica.

si è intervenuti su aspetti obiettivamente secondari, che però hanno finito per dare un contribuito positivo all'impianto stesso del disegno di legge. Il testo all'esame del Senato non è stato modificato in Commissione: sono stati presentati emendamenti relativi alle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, su cui i relatori hanno espresso parere contrario, così come ha fatto anche il Governo. crediamo che sia venuto il momento di approvare finalmente il disegno di legge in esame. È passato circa un anno da quando se ne iniziò l'esame.

Si è parlato lungamente dell'ingresso clandestino; la fattispecie di cui al comma 16 non è stata modificata dalla Camera dei deputati e quindi gli aspetti più delicati che avevano caratterizzato il disegno di legge sicurezza approvato in Consiglio dei ministri non sono stati in alcun modo toccati dalla Camera dei deputati. È per questo motivo che, come relatore, confido in una rapida approvazione del disegno di legge in discussione, che è particolarmente atteso non dai parlamentari della maggioranza, ma dal popolo italiano.

Signor Presidente, torna all'esame del Senato il cosiddetto pacchetto sicurezza, sicurezza, con una serie di modifiche apportate dalla Camera dei deputati, alcune delle quali correttive, e anche positive, altre in realtà più o meno formali. La cosa che più ci preoccupa e che desta particolari motivi di apprensione è che questo provvedimento torna con gli stessi profili di incostituzionalità con cui era stato, ahinoi, licenziato dal Senato.

con le norme e i principi della nostra Carta costituzionale, a cominciare ovviamente dall'introduzione della nuova figura di reato

dei principi di eguaglianza e di tutela dei diritti fondamentali della persona umana. L'errore di fondo che viene compiuto è quello di distinguere, in questo caso, tra la tutela giurisdizionale accordata ai cittadini

e rientra nell'ambito dei diritti della persona. Alle persone che si trovano nel territorio del nostro Stato, e che quindi sono soggette all'amministrazione anche giudiziaria del nostro territorio, conferita una serie di diritti che non possono essere affievoliti da procedure aggravate, speciali e diverse, quelle che vengono introdotte solo ed esclusivamente per questa fattispecie di reato. Il primo aspetto che mettiamo in evidenza è che l'introduzione del reato di soggiorno illegale, di clandestinità, determina sostanzialmente l'adozione di una procedura speciale

Anche a voler ragionare sotto un profilo di natura squisitamente ipotetica sulla circostanza che l'eccezionalità del fenomeno della immigrazione clandestina e delle relative irregolarità sia tale da giustificare una legislazione speciale,

dunque, l'incostituzionalità? Non solo perché viene introdotto un rito speciale senza che ve ne sia la necessità, operando dunque a soli fini discriminatori, ma perché sostanzialmente si utilizza surrettiziamente la classificazione in termini di reato della fattispecie di ingresso e soggiorno illegale per ottenere altri due scopi,

per gli irregolari e, per altro verso, consentire sostanzialmente per di far avvenire in via giudiziale ciò che in via amministrativa è già previsto, ma non funziona bene. Quindi, ci troviamo di fronte all'utilizzo improprio di una norma con un ulteriore effetto negativo, quello dettato dall'allineamento conseguente all'introduzione del reato di immigrazione clandestina con l'articolo 331 del codice di procedura penale, che prevede l'obbligo di denunzia, giustamente, per i pubblici ufficiali e per gli incaricati di pubblico servizio per qualsiasi ipotesi di reato di cui vengano a conoscenza. Ciò sta a significare che l'introduzione del reato di immigrazione clandestina non è funzionale a giudicare in termini di di maggior disvalore sociale quella condotta, ma serve a fare in modo che cambi il sistema di controllo e che porti sostanzialmente all'esclusione da qualsiasi forma di censimento, di accertamento e di rilievo giuridico per gli stranieri irregolari. Questo non aiuta

che prevede l'obbligo per i medici di non denunciare i clandestini e che lo si estenda, sotto forma di non necessità dell'esibizione del titolo di soggiorno, anche alle scuole, quindi all'accesso alle prestazioni scolastiche, non significa nulla, considerato il mantenimento - se resta così, come rimarrà - del reato di immigrazione clandestina. Infatti è evidente che - ad esempio, per quanto riguarda le dichiarazioni relative agli atti dello stato civile dello stato civile - tutta quell'attività che qualsiasi persona che si trova sul territorio dello Stato è tenuta a fare per poter essere conosciuta dall'ordinamento, ivi comprese quindi le variazioni le variazioni residenziali, anagrafiche e quant'altro, è assolutamente inibita allo straniero irregolare: è evidente che l'irregolare che si presenta presso l'ufficiale dell'anagrafe per fare un cambio di residenza determina l'obbligo giuridico da parte dello stesso pubblico ufficiale di denunciarne il reato di clandestinità. Quindi, anche l'iscrizione all'anagrafe dei minori stranieri figli di irregolari è preclusa e tutto questo produce effetti nefasti sotto il profilo della conoscenza del fenomeno della irregolarità da parte dello Stato e degli organi di polizia; d'altro canto, determina altresì l'assoluta invisibilità di centinaia di migliaia di persone e di bambini, in violazione delle convenzioni internazionali che sono a presidio e a tutela dei diritti del fanciullo. Tutto ciò solo per un approccio ideologico che è palesemente in contrasto con i princìpi fondamentali che regolano la nostra Carta costituzionale. Questo è uno degli aspetti, quello più evidente e - se mi è consentito - anche il più ridicolo e paradossale che noi troviamo nel pacchetto sicurezza. Si introduce infatti una nuova figura di reato non per perseguire quella condotta illecita, ma per accelerare procedure amministrative che non funzionano ai fini dell'espulsione e per marginalizzare categorie di soggetti che vanno invece conosciuti, per quello che è possibile integrati e per quello che è possibile respinti al di fuori del territorio nazionale. È un sistema che non tiene, è un sistema illogico e irrazionale, è un sistema che introduce un'inutile disparità di trattamento e una profonda diseguaglianza e che aiuta il circuito dell'illegalità e dell'irregolarità per quanto riguarda gli stranieri. I profili che noi evidenziamo non riguardano solo questo aspetto; ve n'è un secondo - vado rapidamente alle conclusioni - che attiene alle cosiddette ronde.

sono incostituzionali per due ragioni gravi e fondamentali. La prima è che l'articolo 117 della Costituzione attribuisce allo Stato in via esclusiva la competenza in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblici. Sicché, tutti i soggetti che, anche sotto il profilo dell'attività sussidiaria, collaborano con attività che non sono degli enti locali, ma dello Stato (cioè la tutela della sicurezza pubblica), non possono essere oggetto di una disciplina che attribuisce poteri e facoltà ai sindaci. Non possono cioè essere i sindaci a decidere se fare o non fare le ronde e con chi farle, perché deve essere sempre lo Stato, secondo quanto prevede l'articolo 117; i sindaci possono prevederlo solo ed esclusivamente per le attività di supporto legate alla polizia amministrativa locale. Con riferimento alle attività collegate alle competenze della polizia amministrativa locale, le ronde possono essere pertanto utilizzate; per quanto riguarda, però, l'attività di supporto alle forze dell'ordine, non può essere il sindaco a deciderne l'utilizzo, l'impiego e le finalità - ancorché nell'ambito di criteri stabiliti dal Ministero dell'interno - perché l'articolo 117 della Costituzione attribuisce questa competenza in via esclusiva allo Stato

l'articolo 18 della nostra Costituzione prevede espressamente il divieto di autorizzare e costituire associazioni con finalità militari o paramilitari, di carattere più o meno politico. Nel testo al nostro esame, come dimostrano peraltro i fatti di queste ultime settimane, non vi è alcuna disciplina specifica che vieti, in maniera diretta o indiretta, la possibilità che le cosiddette ronde possano essere costituite come strutture paramilitari e politiche di questa o di quella forza. Ci troviamo così di fronte ad una precisa violazione dell'articolo 18 della Costituzione, con tutte le conseguenze che ne discendono. sottolineando che queste disposizioni introducono un sistema che esclude la tutela dei minori non accompagnati nel nostro territorio, costituendo una legislazione speciale in violazione dei diritti fondamentali del fanciullo ed escludendo la possibilità che il neonato possa essere iscritto nei registri dell'anagrafe

Presidente, onorevoli colleghi, signori membri del Governo, il provvedimento all'esame, anche dal punto di vista del Gruppo dell'Italia dei Valori, presenta molteplici aspetti d'incostituzionalità.

Non può costituire argomento giustificativo la previsione della facoltà di arresto da parte di privati, di cui dall'articolo 383 del codice di procedura penale limitata ad alcuni delitti perseguibili d'ufficio, perché è ipotesi eccezionale che non permette di essere allargata. Vi è una perplessità di ordine generale sull'idea delle ronde come corpo specializzato paramilitare

nella norma di «segnalare alle Forze di polizia dello Stato o locali, eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». Mi soffermo un attimo sull'uso del termine «disagio sociale» perché introduce un elemento di indeterminatezza che rispecchia la genericità complessiva del provvedimento. Che vuol dire: «disagio sociale»? Questo termine può avere un senso attivo o passivo; se lo si considera sotto i due profili, appare manifestamente diverso e contrastante. L'idea che la ronda possa giudicare, nell'attività che svolgerà in strada, in merito ad un disagio sociale implica un criterio di conoscenza sociologica e di interpretazione della realtà che sfugge all'immaginazione. Il comma 41 dell'articolo 3 prevede l'iscrizione delle associazioni in questione in un apposito elenco tenuto a cura del prefetto, previa verifica da parte dello stesso, sentito il comitato provinciale per Tale iscrizione non si configura come un'autorizzazione amministrativa, ma come una verifica della corrispondenza tra i requisiti stabiliti nel decreto ministeriale e quelli posseduti dall'associazione. Non si determina un effettivo controllo sull'attività svolta effettivamente dall'associazione. Nel presente disegno che le associazioni non debbano avere né natura né finalità di ordine politico, in considerazione del divieto, posto dall'articolo 18, comma 2 della Costituzione, di costituire associazioni che, anche indirettamente, perseguano scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare in atto la presentazione al pubblico di ronde che si autorappresentano attraverso uniformi. Si profila un'organizzazione di tipo gerarchico, che ha un'analogia con l'organizzazione militare e che è rafforzata dall'uniforme. Si potrebbe persino ironizzare sugli stilisti delle uniformi che si stanno già manifestando sulla scena.

ronde a soggetti che sono stati condannati per reati di violenza o compimento di atti di discriminazione per motivi razziali, etnici o religiosi. La convinzione è che la genericità delle previsioni relative alla configurazione complessiva delle ronde, contenuta in questo disegno di legge, potrà più facilmente incrementare il rischio di incidenti, piuttosto che sollevare il compito delle forze dell'ordine. Molto più prevedibilmente costituirà un aggravio del lavoro delle forze dell'ordine perché le distoglierà dai compiti effettivamente loro

di forte criticità relativo a questo provvedimento riguarda la questione dell'ingresso e del soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Con la disposizione di cui al comma 16 dell'articolo 1 diventa reato non solo l'ingresso illegale, ma anche la permanenza sul territorio. Tale misura è incompatibile con l'articolo 24 della Costituzione. La norma si presta ad una pluralità di osservazioni critiche che hanno, come punto di partenza, la constatazione dell'eccezionale aggravio che la sua introduzione comporterebbe per l'attività giudiziaria in generale. in generale. Una contravvenzione punita con una pena pecuniaria non appare prevedibilmente efficace per chi è spinto ad emigrare da condizioni disperate.

Né il provvedimento appare idoneo a conseguire l'intento di evitare la circolazione nel nostro Paese di stranieri entrati irregolarmente, poiché già la normativa vigente, in base al combinato disposto degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 25 n. 286, consente alle autorità amministrative competenti di disporre l'immediata espulsione. Di fronte a questo, pare ragionevole la previsione di un aggravio per l'amministrazione della giustizia.

che chiede di contrarre matrimonio in Italia. Si preclude direttamente la possibilità di creare una famiglia e quindi si rende più difficile la possibilità dell'integrazione, in palese violazione dell'articolo 29 della Costituzione.

criticità - dispone di estendere a 180 giorni il periodo massimo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione.

perché il comportamento dell'immigrato potrebbe essere vincolato sia alla propria volontà di mantenersi nella sua condizione sia all'incapacità dello Stato di

dell'intervento: la resistenza all'identificazione legittima il trattenimento, i ritardi nell'ottenimento della documentazione legittimano solo il prolungamento della permanenza», Inoltre, la attribuzione della competenza relativa alla proroga del trattenimento attribuita al giudice di pace è anomala perché si tratta di provvedimento che è inerente alla materia della privazione della libertà personale e appare fuori luogo attribuire il carico di un argomento di così vitale importanza

Ci sono altri elementi di irragionevolezza e indeterminatezza e questi contrastano con il criterio di ragionevolezza delineato dall'articolo 3

La lettera *t)* del comma 22 dell'articolo 1 sembra arrivare ad impedire il ricongiungimento del genitore naturale con il minore, nel caso in cui l'altro genitore sia deceduto o sconosciuto. Tutti questi elementi concorrono a determinare un quadro in cui appare fondamentale, nella logica del provvedimento,

proclamato dalla Costituzione repubblicana e quindi, in base a questo, il Gruppo dell'Italia dei Valori oppone il suo più fermo giudizio contrario.

non possa essere effettuata alcuna operazione di voto sulle questioni stesse. Tale voto avverrà nella seduta antimeridiana di domani.

La Presidenza non si sarebbe concessa questa gratuità per accontentare la maggioranza e liberare l'Aula. La Presidenza si è fatta carico di realizzare le opportune intese con tutti i Gruppi, senatrice Poretti.

del disegno di legge che noi ci apprestiamo ad approvare introduce nell'ordinamento il reato di immigrazione clandestina e permanenza illegale, a titolo di reato contravvenzionale, ossia è punito non solo l'ingresso irregolare ma anche il soggiorno illegale nel territorio dello Stato. I commi da 30 a 32 dell'articolo 1, si preoccupano di quantificare gli oneri recati

Ovviamente, la quantificazione dei costi e quindi la necessaria copertura finanziaria per questa duplice fattispecie di reato deve essere rapportata alla platea dei destinatari della norma. Originariamente, come lei, signor Presidente, e gli altri colleghi ricorderanno, l'ipotesi di reato era quella di ingresso illegale e si quantificavano in 54.000 gli ingressi illegali annui nel nostro Paese, sulla base dei dati statistici degli anni precedenti. Si assumeva che l'effetto dissuasivo della norma - ma la sanzione all'epoca era quella della reclusione da sei mesi a quattro anni,

nella relazione tecnica, ha stimato che ogni processo avrebbe avuto un costo di 650 euro, determinato dal gratuito patrocinio, dall'interprete e accessori vari. Quindi, moltiplicando 650 euro per 49.050, ossia il numero dei destinatari della norma, si arrivava alla copertura di 33 milioni di euro.

dati forniti dal Ministero dell'interno per assumere la congruità della copertura finanziaria indicano... RUSSO *(IdV)*. Presidente, Presidente,

Allora, la relazione tecnica assume...

Il Ministero dell'interno ha stimato e ha dichiarato nella relazione tecnica

dei soggiornanti illegalmente nel nostro Paese è di 3.660 persone, e questo è un falso!

che gli stranieri irregolari nel nostro Paese sono 760.000. In base a quale documento il Ministero dell'interno ha potuto fornire il dato falso, secondo cui

comporta oneri connessi al patrocinio a spese dello Stato quantificabili in relazione alla platea degli imputati astrattamente interessati,

quelli relativi al numero di soggiorni irregolari sono stati comunicati dal Ministero dell'interno-Dipartimento della pubblica sicurezza;

Come fa il Ministero dell'interno a parlare di 3.660? Si è detto un falso per giustificare una inadeguatissima copertura finanziaria, stimata in 33 milioni di euro, mentre ci vogliono 600 milioni di euro, ossia 650 euro, quanto secondo il Ministero viene a costare ogni singolo processo, Rispondete allora con chiarezza su questo punto. L'ho sollevato in Commissione, e il sottosegretario Mantovano non ha voluto rispondere. Ho reiterato la richiesta in Commissione: silenzio assoluto. Lo pongo in quest'Aula, perché vi

*(PD)*. Signora Presidente, signori del Governo, signori senatori, sono diverse le disposizioni di questo provvedimento che generano rilevanti perplessità, sia di ordine costituzionale, sia di ordine politico. Non è un caso che in prima lettura in quest'Aula il Governo sia stato battuto per ben tre volte: questo è stato un segno dei forti contrasti all'interno della maggioranza sulle norme che riguardano le cosiddette ronde, i centri di identificazione e di espulsione e le norme in materia di immigrazione. È un segno, questo, della pericolosità di alcune norme che sono state approvate alla Camera dei deputati e che ci vengono riproposte in quest'Aula. Non è un caso che, proprio per superare questi forti contrasti all'interno della maggioranza, presso la Camera dei deputati siano stati imposti - sottolineo: così come si parla anche quest'oggi della imposizione del voto di fiducia in Senato, anche per l'ulteriore passaggio di questo disegno di legge, esclusivamente per problemi vostri, per problemi di questa maggioranza. Viene quasi da parlare di voti di scambio, proprio per questo scambio di voti di fiducia. La Lega Nord che cede sulle intercettazioni telefoniche e da parte sua, il PdL, per non essere da meno, che cede in tema di sicurezza. Ma di quale sicurezza state parlando? Qual è davvero la vostra priorità? Mentre voi parlate teoricamente di lotta alla criminalità, presentate in Commissione giustizia di questo Senato - e ne stiamo discutendo da oggi - di un disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche che è un disegno di legge criminale, perché favorisce i delinquenti, i criminali *(Applausi dal Gruppo PD)* ed è un disegno di legge liberticida nei confronti della libertà di stampa. E ora decidetevi, signori del Governo e della maggioranza: chi volete tutelare? I delinquenti o i cittadini? E ora ci venite a proporre con questo disegno di legge l'istituzione delle cosiddette ronde. Propaganda. È soltanto propaganda. Credo che qualcuno, dai banchi del Governo e della maggioranza, non si sia reso conto, non si renda conto a che cosa si sia data la stura. Basta leggere le cronache di queste ultime settimane: si è parlato di "ronde nere" a proposito di quell'associazione milanese che aveva dotato i propri associati di materiale e di divise di stampo militaresco e di emblemi nazifascisti; si è temuta la costituzione, in certe zone dell'Italia del Sud, di gruppi di cittadini assoldati dalla criminalità organizzata; ci sono stati scontri a Padova tra ronde padane ed esponenti dei centri sociali;

È successo, sempre in questi giorni, addirittura che si siano verificati scontri e accuse pesanti tra due Ministri di questo Governo e assessori della Giunta regionale

abbiamo i poliziotti, sempre più spesso chiamati a far da guardia, anche nottetempo, alle ronde, per evitare che queste combinino guai o creino disordini: vengono così distolti dai loro compiti istituzionali. Ma invece di far perdere tempo alla Polizia e ai Carabinieri, signori del Governo, pensate piuttosto di dotarli di mezzi e strumenti per operare al meglio! Stanziate risorse finanziarie pari almeno alle tante vostre parole! *(Applausi dal Gruppo PD).* Guardate, signori del Governo e della maggioranza, che in fase di prima lettura abbiamo già evitato un grosso rischio. Ricordo che inizialmente il testo del vostro disegno di legge parlava *sic et simpliciter* di ronde, senza vietare l'uso di armi e con compiti anche di presidio del territorio. Di fronte alla nostra preoccupata segnalazione di pericolo sociale ed istituzionale che ciò comportava, in Commissioni 1a e 2a riunite, Governo e maggioranza ci hanno risposto picche: hanno approvato ronde tacitamente armate con compiti di presidio del territorio. Una cosa istituzionalmente da pazzi, perché venivano così legittimate bande armate paramilitari sul territorio, dell'uno o dell'altro partito, dell'una o dell'altra organizzazione criminale, in spregio anche all'articolo 18 della Costituzione. Per buona sorte, in occasione del primo passaggio in Aula del Senato, per resipiscenza del Governo e per lucida tenacia dell'opposizione, il peggio veniva scongiurato. Ora però la cronaca, i duri fatti ci danno ragione anche sulla parte restante delle nostre critiche. I duri fatti vengono a confermare tutte le nostre preoccupazioni. badate bene che a legislazione vigente i sindaci e le varie amministrazioni locali sarebbero e sono benissimo in grado di intervenire a tutela dei cittadini: l'esperienza dei Comuni di Milano, Bologna, Padova ed altri Comuni del Veneto lo sta a confermare. Invece, le norme sulle cosiddette ronde che si dovrebbero approvare stravolgono il tessuto istituzionale e costituzionale e, non a caso, sono fortemente contestate anche dagli operatori della sicurezza, proprio per la loro pericolosità. Le norme odierne rischiano di assegnare a privati la titolarità di funzioni in un ambito, quale quello della gestione dell'ordine pubblico e della tutela della pubblica sicurezza, che costituisce un'attribuzione tipica ed esclusiva dell'istituzione statuale, proprio perché tali delicatissime funzioni a garanzia dell'incolumità e della libertà di tutti devono essere esercitate nel pieno rispetto della legge e con il massimo grado di imparzialità, professionalità, proporzionalità ed adeguatezza e nel rispetto dei diritti dei cittadini che solo l'autorità di pubblica sicurezza può pienamente garantire. Le norme oggi in esame sono chiaramente incompatibili con il principio del nostro ordinamento che assegna allo Stato il monopolio della forza, affinché questa venga esercitata nelle forme previste dalla Costituzione e dalla legge, a tutela dell'incolumità e della sicurezza delle persone e nel rispetto della dignità della persona, dell'uguaglianza dei diritti e delle libertà di tutti. Si tratta di un principio generale dell'ordinamento che trova esplicito riconoscimento nel testo costituzionale, che autorizza soltanto la pubblica autorità all'utilizzo legittimo di ogni forza di coercizione fisica. Infine, ricordo come le norme di cui ai commi 40 e seguenti dell'articolo 3 non sanciscano espressamente il carattere non violento di tali associazioni ma solo il fatto che quanti ne fanno parte non siano armati. Nulla esclude perciò, come in qualche caso è già successo, che le cosiddette ronde, magari perché ispirate ad opposte ideologie politiche, possano venire alle mani o che talune di esse possano compiere atti squadristi di aggressione o di mortificazione nei confronti di soggetti ad esse invisi, come, per esempio, gli immigrati, e che la loro stessa esistenza possa essere interpretata come un segno di debolezza delle forze di polizia e finisca per generare sfiducia nelle istituzioni; che insomma queste cosiddette ronde si trasformino in fattori di insicurezza e disordine pubblico, alla faccia della da voi tanto conclamata esigenza di sicurezza. Per queste considerazioni, chiediamo che il Senato deliberi di non procedere all'esame delle norme del disegno di legge n. Presidente, il suggerimento che la coscienza fornirebbe sarebbe quello di manifestare ancora una volta indignazione per molte delle norme contenute nel testo di legge sul quale alcune

numeroso", ci si debba attenere alle questioni tecniche di cui la tematica in discorso è costellata. In particolare, mi occuperò di una questione pregiudiziale di costituzionalità dell'articolo 1, comma 22, lettera *l)*, del testo di cui parliamo. Tale norma dispone l'estensione del termine massimo del trattenimento dello straniero nei centri per l'identificazione e l'espulsione da due a sei mesi si tratta di una durata di detenzione sostanziale comminata, nella sostanza dei fatti, anche per reati di cospicua gravità, come ad esempio il furto aggravato) aggravato) per i casi di mancata cooperazione al rimpatrio del Paese terzo interessato o ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi. In proposito, è stata evocata a sostegno di tale impostazione la direttiva comunitaria

di ipotesi di riduzione della libertà personale caratterizzate dal principio di proporzionalità. Il punto 16 dei considerando della direttiva in discorso afferma infatti testualmente che «il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi adottati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento è giustificato soltanto per preparare il rimpatrio o effettuare l'allontanamento e se l'uso di misure meno coercitive è insufficiente». In maniera implicita, ma fortissima, tale disposizione allude alla necessità di una graduazione di misure e alla predisposizione anche di misure meno coercitive, di cui non vi è traccia nel provvedimento oggi in esame. L'articolo 15 della direttiva in questione dispone inoltre il ricorso al trattenimento solo nei casi in cui non possono «essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive» e precisa altresì

preparazione del rimpatrio o dell'allontanamento» (che è un concetto ben diverso da quello di mancata cooperazione, come sa bene chiunque abbia una qualche dimestichezza con le norme). La norma in esame non prevede alcuna misura alternativa alla detenzione, la quale resta di fatto l'unica misura prevista, senza che sia possibile valutare l'efficacia e la sufficienza di misure meno coercitive. Infine, questa norma, disponendo la possibile estensione a centottanta giorni del periodo di trattenimento, determina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione (questo è il punto tecnico della questione pregiudiziale), una irragionevole discriminazione fra stranieri di provenienza diversa, poiché stabilisce che la durata maggiore o minore della detenzione sia di fatto condizionata arbitrariamente dalla maggiore o minore efficienza burocratica dei diversi Paesi di origine. Pertanto, un cittadino di Stato terzo proveniente da un Paese maggiormente arretrato potrebbe subire, solo a causa a causa di questa condizione, una detenzione pari ad un tempo superiore del doppio ed in alcuni casi addirittura del triplo rispetto a quello ordinariamente stabilito. e per il chiaro contrasto con la disposizione dell'articolo 3 della Costituzione, che noi chiediamo che il Senato non proceda all'esame del disegno di legge n. 733-B.

credo sia opportuno ricordare, ancora una volta, il modo di lavorare di questa Assemblea. L'annuncio effettuato dal presidente Schifani, che poi si è allontanato, è del tutto legittimo; però, esso determina lo svuotamento dell'Aula: anche questo è legittimo, ma è evidentemente un piccolo ulteriore passo verso lo svuotamento dell'attività democratica dell'Assemblea. Lei pure, signora Presidente, è poco interessata a quanto sto dicendo: mi segua. La questione pregiudiziale QP6 al disegno di legge in esame si riferisce in particolare all'articolo 1, Esso subordina il rilascio (e il rinnovo) del permesso di soggiorno alla stipula di un "accordo di integrazione" tra straniero e Stato, in cui il primo si impegna a conseguire obiettivi di integrazione non meglio specificati.

Tale imprescindibile prescrizione dovrà essere definita da un regolamento. Vedremo appresso quali saranno gli effetti normativi del ricorso a questo strumento. articolo 1 dispone che la perdita integrale dei crediti determina l'espulsione immediata dello straniero, peraltro non sospendibile neppure qualora egli ricorra in giudizio avverso il provvedimento espulsivo.

si intende con integrazione quel processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto dei valori sanciti dalla Costituzione italiana, con il reciproco impegno a partecipare alla vita economica, sociale e culturale della società». Ebbene, colleghi (mi rivolgo a quelli interessati), vi sembra logico che il perseguimento di tali obiettivi sia posto a carico del povero straniero che stipula l'accordo e si impegna a rispettare In caso di mancato rispetto o mancata realizzazione di questi alti obiettivi, da ogni punto di vista, ne consegue l'espulsione e non è neppure dato sapere se l'espulsione seguirà per fatto colpevole o incolpevole.

nella misura in cui esso limita la facoltà (giammai l'obbligo) degli Stati di subordinare alla verifica dell'integrazione dello straniero la sola concessione del permesso di soggiorno per lungo periodo. Nel periodo lungo ha un senso parlare di integrazione,

Al contrario, si evince che, in relazione alla concessione del permesso di soggiorno ordinario, non è in facoltà degli Stati subordinare tale diritto soggettivo ad una situazione come quella dell'avvenuta integrazione, tanto più che tale situazione non dipende, se non in minima parte, dalla volontà e dal comportamento del soggetto istante. Ciò sfugge al legislatore o alla maggioranza. E, che si tratti di un diritto soggettivo dell'istante, lo si evince dalla incontestabile circostanza che la legittima aspettativa dell'immigrato a poter soggiornare in uno Stato trova la sua più forte e profonda legittimazione nel diritto naturale, che riconosce ad ogni persona il diritto a trasferirsi, per ragioni non certo illecite, ma addirittura in ragione di un'impellente necessità (quale può essere la fame o la guerra, che generalmente caratterizzano le motivazioni di un'onda così immane dal punto di vista storico della migrazione che stiamo vivendo), da un territorio all'altro e da uno Stato ad un altro. Tale assunto sembra trovare conforto, nel nostro sistema, anche nelle decisioni della Corte costituzionale, che in alcuni provvedimenti in materia propende infatti per la qualificazione di diritto soggettivo e non per quella di interesse legittimo *tout court*, con la conseguenza di una impossibilità, per l'autorità amministrativa, a condizionare il riconoscimento di tale diritto alla sussistenza della dimostrazione dell'avvenuta integrazione del migrante,

alla valutazione (necessariamente discrezionale), da parte dell'autorità amministrativa, del grado di integrazione del soggetto. È infatti evidente che l'integrazione costituisce un percorso complesso, che nessuna autorità amministrativa potrebbe giudicare con precisione se non fornendo pareri del tutto arbitrari e quindi inevitabilmente discriminatori. A ciò si aggiunga che la legge non stabilisce né il criterio sulla cui base tale valutazione deve condursi, né quali fatti determineranno la perdita dei crediti, ma rinvia tutto ad un regolamento governativo: lascia dunque che sia una fonte secondaria a normare un diritto soggettivo. Ciò comporta una palese violazione dell'articolo 10, secondo comma, della Costituzione, che sancisce una riserva di legge (peraltro rinforzata) in materia di disciplina della condizione giuridica dello straniero. è evidente che tale riserva non è soddisfatta se la disciplina effettiva della condizione dello straniero (gli atti che determinano la perdita dei crediti, i criteri di valutazione dell'integrazione e così via) è rimessa integralmente alla fonte regolamentare. la norma appare contrastare con il diritto internazionale e con la protezione accordata dall'articolo 10 della Costituzione agli asilanti, nella misura in cui non esclude - questo è un aspetto importantissimo - dalla possibilità di espulsione i titolari di protezione umanitaria, i rifugiati e gli asilanti. Del tutto irrilevante appare la circostanza che attiene alla persistente mancanza nel nostro Paese di una normativa precisa, completa ed adeguata in merito al diritto di asilo. Resta infatti indiscutibile la natura del diritto soggettivo all'asilo, come riconosciuto dalla Costituzione, così che l'entrata in vigore della norma in discussione comporterebbe, e comporterà, una evidente violazione dell'articolo 10 della nostra Costituzione, impedendo in questi casi completamente - come si sta ampiamente verificando: è sufficiente pensare al respingimento dei barconi in Libia - 1'esercizio del diritto di asilo a coloro che ne potrebbero beneficiare. Per queste ragioni, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 733-B in esame.

ma direi anche gravi dal punto di vista della civiltà, non solo giuridica, ma dei comportamenti di un Paese e di una Nazione civile. In particolare, il citato articolo 6, comma 2, nel precedente testo, prevedeva che, per quanto concerne i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e gli atti di stato civile o l'accesso ai pubblici servizi,

questo premesso. Questo comma è stato modificato: il risultato è che per rivolgersi agli uffici dello stato civile, e quindi per avere i servizi relativi, o per accedere ai pubblici servizi bisogna avere ed esibire il permesso di soggiorno, fatte salve, si dice, le prestazioni sanitarie - sappiamo anche quante polemiche sono state fatte in proposito, con vari cambiamenti - e le prestazioni scolastiche obbligatorie. È evidente che questo tipo di previsione contrasta con la nostra Costituzione in molti suoi aspetti e con le convenzioni internazionali, in particolare con quella dell'ONU per quanto riguarda i diritti dell'adolescenza. Ci troviamo di fronte ad alcuni paradossi, giuridici e civili: la violazione degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, relativi ad esempio al diritto di contrarre matrimonio, al dovere dei genitori di mantenere i figli

e con tutte le previsioni che ho citato, nonché, appunto, con molte convenzioni internazionali. Ma io mi domando: se la sicurezza è - e lo è davvero - una delle preoccupazioni testa dei nostri cittadini, se è una questione di rilevanza nazionale e internazionale sulla quale è giusto intervenire e dare risposte adeguate alla complessità dei fenomeni, e se questi fenomeni hanno una dimensione sociale, politica e geopolitica molto complessa, la risposta può davvero essere questa? Può essere quella di vietare ad una donna, in realtà in modo molto chiaro e netto, anche se non dal punto di vista della previsione giuridica, di partorire in un ospedale perché non sa quale fine farà il proprio figlio, perché non può dichiararlo, perché probabilmente verrà strappato ai genitori, alla madre e al padre, perché suo figlio sarà - come è stato detto - un figlio invisibile? Che c'entra questo con il contrasto ai fenomeni della clandestinità? Che c'entra questo con il governo dei flussi migratori? Quale Paese civile pensa di arrivare a queste aberrazioni giuridiche e sociali? Credo che dovremmo riflettere molto approfonditamente, perché la complessità di questi fenomeni non ha mai trovato il Partito Democratico in un atteggiamento minimalista o riduttivo nel voler affrontare, governare e anche contrastare alcuni aspetti degli stessi. Ma noi non possiamo trovarci di fronte a questi paradossi. L'impossibilità di contrarre matrimonio, come tutti sanno, è un elemento non relativo alla cittadinanza ma che riguarda i diritti fondamentali; non possiamo trovarci di fronte a questa violazione che riguarda le persone, gli esseri umani, al di là di ogni politica di contrasto sulla quale pure abbiamo espresso, con i nostri emendamenti, delle posizioni molto ferme, dando un contributo anche in questa direzione. direzione. Su questi temi un Paese civile trova la strada per unire sicurezza e diritti; trova la strada per governare fenomeni complessi. La prima strada avrebbe dovuto essere quella di rivedere la legge Bossi-Fini, per la quale migliaia e migliaia di questi bambini, di queste donne, di questi uomini possono trovarsi esposti continuamente alla precarietà della loro vita e del loro futuro, perché da un momento all'altro, con la scadenza del permesso di soggiorno, diventano clandestini. Immaginate quale sicurezza potranno avere questi bambini, quale prospettiva per il futuro della loro vita, della loro salute; pensate quali pregiudizi possiamo creare ad esseri umani verso i quali un Paese civile è obbligato a dare risposte, pur se deve affrontare con una mano ferma, dal punto di vista dei temi che riguardano la clandestinità, i fenomeni connessi criminali: sicuramente con una mano ferma, dando un aiuto alle forze dell'ordine. Ma voi non avete fatto altro che sbandierare paure e mettere in campo ricette che sono inefficaci, addirittura inutili e molto spesso dannose; dannose dal punto di vista giuridico per l'ambiguità e la violazione dei diritti. Pensate che questa nuova formulazione così ambigua che non si capisce per esempio nemmeno, quando si muore, se si potrà andare a dichiarare la morte presso lo stato civile se non si ha il permesso di soggiorno; pensate a quale aberrazione giuridica e della vita reale state portando molti territori che sono pieni di queste presenze, e pensate cosa state facendo a tanti bambini, a tante donne, a tante famiglie. Questo è davvero molto grave. L'Italia è un Paese civile. Oggi nel mondo 50 milioni di bambini non sono registrati: fanno parte dei Paesi sottosviluppati. Cosa vogliamo fare come Paese civile? Metterci sulla stessa strada? Credo che, per le ragioni che ho esposto, per i motivi e le complessità che sono legati a questi fenomeni, la strada avrebbe dovuto essere tutt'altra: quella di rivedere la legge, quella, sicuramente, di soffermarsi sul governo di questi fenomeni, ma non quella di cercare scorciatoie aberranti dal punto di vista sociale e giuridico. A nulla sono valsi gli appelli e i documenti di tantissime associazioni, dai salesiani alle ACLI, alle associazioni giuridiche, così tante che non si possono nemmeno qui elencare per ragioni di tempo; non sono valsi a niente. Questo Governo non ha fatto altro che sbandierare paure e trovare soluzioni ancora più misere di queste stesse paure. È per questo che siamo nettamente contrari

un fronte di riflessione che non potrà essere discusso, ma forse può essere l'inizio di una riflessione comune, per l'inopinata decisione del Governo - ormai risulta - di porre la fiducia; la fiducia, peraltro (va detto), non tanto perché gli emendamenti fossero molti o perché ci fosse chissà quale problema, ma più modestamente - si fa per dire perché la possibilità di voti segreti, a norma di Regolamento, per quanto riguarda articoli ed emendamenti di aderenza costituzionale, evidentemente non rassicurava abbastanza la maggioranza.

Mi riferisco ai circa 500.000 immigrati nel nostro Paese, irregolari perché non in possesso di tutti i documenti, che però, in base alla legge Bossi-Fini, hanno fatto «la coda» per depositare tutti i documenti richiesti. Questo significa che le nostre autorità

il flusso ne ha autorizzati 140.000 e 70.000 richieste sono state respinte; rimangono quindi nel limbo totale, presenti sul nostro territorio - anzi, nelle nostre case circa 500.000 fra badanti, colf o, nelle piccole e medie imprese, lavoratori dell'edilizia o dell'agricoltura, che al passaggio di questa legge, oltre che essere irregolari, saranno evidentemente oggetto e vittime del reato di clandestinità. Ma c'è più di questo: il problema è che anche 500.000 italiani (famiglie o datori di lavoro)

centinaia di migliaia di famiglie nel nostro Paese ospitano a casa *babysitter* o badanti; queste *babysitter* o badanti non sono in regola, per le ragioni che ho appena detto. queste persone non osano più uscire di casa: certo non portano i ragazzi a scuola con la macchina, fosse mai che succeda qualcosa, perché non hanno né l'assicurazione né i documenti in ordine; non portano più l'anziano a fare le analisi all'ospedale, per lo stesso motivo; e non vanno a fare la spesa; insomma, vivono chiuse in casa.

È una legge che implica un'applicazione discrezionale; il problema, però, è cosa accadrebbe mettendo fuorilegge una tale massa

compiuto da un Governo e da una maggioranza che, invece, si muovono nell'ottica di rafforzare lo Stato di diritto, convinta come sono - e come penso molti di voi - che l'affermazione della legalità sia uno degli strumenti più potenti

che contribuisce al messaggio dato in tutti questi mesi all'immaginario collettivo, che è il seguente: immigrato uguale crimine, uguale insicurezza, uguale delinquenza.

senza i quali grandi settori del nostro Paese affronterebbero sicuramente una condizione economica piuttosto grave; purtroppo, il messaggio è unidimensionale.

se porrete la fiducia, ma mi auguro che il Governo individui d'urgenza qualche strumento per non negare la possibilità ai cittadini italiani di essere dei buoni cittadini, assieme a quei lavoratori che non hanno passaporto italiano.

il mio compito è quello di illustrare una questione specifica che si riferisce all'impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico esercizi, presente nei commi da 7 a 13 dell'articolo 3 del disegno di legge. Prima però di arrivare all'illustrazione di questa specifica ragione di incostituzionalità, voglio riprendere alcuni degli argomenti che sono stati anche di recente sollevati dalle colleghe Incostante e Bonino, che riguardano, più in generale, il tema di questo disegno di legge, perché mi paiono particolarmente rilevanti. Entrambe le colleghe hanno fatto riferimento alla abnormità dell'introduzione del reato di immigrazione clandestina. La collega Bonino ora si riferiva agli effetti perversi che questo produce, in modo particolare per quelle famiglie che hanno presso di sé delle persone addette alla cura della famiglia stessa in condizioni di irregolarità.

ovviamente in condizione di irregolarità; poi si fa la fila per cercare di essere regolarizzati. Questa è la situazione attuale, voluta da una legge ipocrita, che vuole nascondere l'esistenza di un fenomeno che ormai è costitutivo di tutte le società avanzate, compresa la nostra, fenomeno aggravato, tanto da farne un vero e proprio reato, da questo disegno di legge. ha degli aspetti davvero paradossali e fortemente incostituzionali, perché, come è stato ricordato, produce una serie di effetti a cascata

caccia della badante irregolare per verificare se essa abbia o meno le caratteristiche per stare in Italia regolarmente e quindi eventualmente essere incriminata e multata perché irregolare e clandestina. Pertanto, gli effetti

si è riferito ad un altro aspetto molto evidente di incostituzionalità di questo provvedimento, quello relativo alle cosiddette ronde. Non c'è dubbio alcuno che c'è un principio generale del nostro ordinamento in base al quale l'uso legittimo della forza, con possibilità di costrizione personale, è riservato

funzioni di questo genere, siamo di fronte ad un provvedimento contrario ai principi generali dell'ordinamento e, in modo particolare, all'articolo 13 della Costituzione, che stabilisce per l'appunto il principio secondo il quale l'utilizzo legittimo di ogni forma di coercizione fisica è dello Stato e solo dello Stato. Sulla materia sono state richiamate una legge della regione Emilia-Romagna

né la legge della regione Emilia-Romagna né le esperienze di questi comuni assegnano a soggetti diversi dalle forze dell'ordine il compito di intervenire in materia di tutela dell'ordine pubblico. Invece con questo provvedimento si estende questa possibilità e si viola quindi un principio costituzionale. Concludo illustrando specificamente la ragione della pregiudiziale di incostituzionalità. Ho fatto riferimento ad una declinazione apparentemente minore ma ugualmente molto pericolosa del principio delle ronde, tanto è vero che è stato chiamato in gergo "delle rondìne". Cioè, il fatto che sia possibile nei locali pubblici o aperti al pubblico assegnare, per l'appunto, ad un determinato personale il compito di tutelare l'incolumità dei presenti. Apparentemente si tratta di una norma di buon senso, ma caso bisogna ricordare che tale funzione non viene svolta neanche dalle guardie giurate, che si limitano ad altro tipo di funzione;

da 7 a 13 dell'articolo 3 si viola, invece, un principio generale dell'ordinamento, assegnando a queste persone un compito che è chiaramente di sicurezza pubblica, andando in aperto e chiaro contrasto con l'articolo 13 della Costituzione. signori del Governo e signori della maggioranza, che questo produrrà maggior tutela della sicurezza, maggiore tutela della quiete pubblica con riferimento che comunque debbono essere sicuramente normate perché possono essere fonte di disturbo della convivenza civile? Noi pensiamo di no, perché pensiamo che gli effetti perversi di questa norma e di questo provvedimento saranno tali da violare un principio generale di legalità, che andrebbe invece rigorosamente salvaguardato. Questa è la ragione per cui chiediamo di non procedere al nostro esame, perché ci sono ragioni evidenti di incostituzionalità, tra le quali quelle che ho appena cercato di illustrare.

portando a lettura definitiva, cioè il prolungamento dei termini di permanenza nei CIE,

tutto inaccettabili, sia ad una lettura di merito, sia ad una lettura costituzionale del sistema di accertamento della identificazione dello straniero che arriva in maniera irregolare nel nostro Paese. sottolineare che dietro alcune motivazioni tecniche, che mi appresto ad accennare e che sono a base della pregiudiziale, dietro pregiudiziale, dietro la volontà del Governo di ritornare sul tema vi è una concezione del Parlamento che ci permettiamo di sottoporvi come una concezione negativa e che cancella alcune delle prerogative di libertà del Parlamento. Quando il Governo ha proposto l'allungamento dei termini di permanenza nei CIE e la loro trasformazione da sistemi di identificazione a sistemi di identificazione ed espulsione,

Ha detto un no a voto segreto, ritenendo che la condizione di questi stranieri fosse una condizione che atteneva lo stato di persona e, quindi, profili di libertà della persona umana che debbono essere tutelati non solo ai cittadini ma alla persona, secondo una particolare lettura della nostra Costituzione che in queste Aule è la versione corrente.

cioè come trattare lo straniero, di cui dobbiamo accertare l'identità, la nazionalità, lo *status*, per cercare di capire se vuole entrare clandestinamente nel nostro molto diversamente, può accampare i diritti che le norme internazionali accordano a tutte le persone umane. Ebbene, la maggioranza ed il Governo,

Il Governo vuole moltiplicare i centri di identificazione e di espulsione, finanziandoli con somme - che andrebbero invece meglio destinate ad altre finalità

a meno di non immaginare che nei centri di identificazione e di espulsione si continui a non garantire certi standard di servizi alle persone, mantenendoli assolutamente insufficienti. Mi riferisco in particolare all'assistenza sanitaria e psicologica, al servizio di di orientamento e di assistenza legale - laddove la domanda dello straniero serve a verificare, per esempio, il suo *status* di rifugiato - alla qualità e al numero degli interpreti mediatori, alla qualità, insufficiente, dello standard logistico offerto (si vogliono creare 3.400 posti in più, con circa 30 milioni di euro).

dai tecnici diritto penale dello straniero. Secondo noi, tutto ciò è oltre la previsione della nostra Costituzione, è oltre il dettato della direttiva comunitaria n. che «il ricorso al trattenimento ai fini dell'allontanamento dovrebbe essere limitato e subordinato al rispetto del principio di proporzionalità con riguardo ai mezzi adottati e agli obiettivi perseguiti. Il trattenimento

l'uso di misure meno coercitive non è assolutamente previsto; è prevista semplicemente una sorta di livella, che equipara donne e bambini, minori e persone inoffensive con persone che invece, anche ad una valutazione delle forze di polizia, potrebbero necessitare un diverso trattamento. Facciamo poi dipendere quella che sostanzialmente è una detenzione - e qui in violazione dell'articolo 3 della Costituzione - semplicemente dall'efficienza dei sistemi amministrativi

(o quella che viene definita, in maniera del tutto inopinata e ipocrita, ospitalità nei centri, e che in realtà è una detenzione),

dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, chiediamo di non procedere alla discussione del disegno di legge n.

Signor Presidente, devo dire che vorrei agganciarmi al discorso fatto da altri colleghi e innanzitutto prendere atto, ancora una volta, dell'inutilità del Parlamento: in questo il Presidente del Consiglio ha perfettamente ragione. Abbiamo oggi il Presidente del Senato rappresentato dal Vice Presidente di opposizione e sono, per carità di Patria, presenti in Aula pochissime persone, tra cui il Sottosegretario alla giustizia, mio collega, vincolato al suo posto, e uno dei relatori. Chiaramente, l'annunzio dato dal Presidente del Senato che non si votava ha determinato la possibilità di lasciare immediatamente l'Aula, per cui tutte le questioni di costituzionalità che possiamo sollevare sono assolutamente inutili, sono un discorso tra pochi eletti che condividono soprattutto una conoscenza giuridica più che una conoscenza sociale, che a quanto pare non interessa ad alcuno. Anzi, mi pare di capire che in una situazione di questo genere genere la maggioranza, se dovrà votare la fiducia e la voterà ciecamente, non ha alcun interesse a sentire, perché non lo vuole, se ci sono argomenti per cui il provvedimento che si accinge ad approvare è incostituzionale. Noi peraltro siamo qui non soltanto perché siamo opposizione, ma perché crediamo seriamente che questo provvedimento, passato già all'esame del Senato e della Camera, sia incostituzionale e lo dobbiamo dire perché non possiamo ingannare i cittadini italiani in merito alla sicurezza. Esso è incostituzionale sotto vari aspetti e mi colpisce sinceramente che ormai questo nostro sistema politico, come esattamente dice Stefano Rodotà, viva quotidianamente ai margini della legalità costituzionale, alterando il funzionamento del sistema istituzionale, che poi finisce con il trasferire il compito di garantire un corretto funzionamento del sistema stesso ad alcuni custodi: il Presidente della Repubblica, la Corte Costituzionale di cui si accentua invece la politicità e l'inadeguatezza e - e - orrore! - il giudice ordinario, quel giudice ordinario che in realtà non si vorrebbe in alcun modo farlo funzionare e con questo provvedimento si fa di tutto per non farlo funzionare. se c'è una prima violazione della norma costituzionale è quella dei tempi del processo. Il giusto processo sancito dall'articolo 111 della Costituzione, con questo provvedimento va a farsi benedire. della giustizia, che giustamente il senatore Li Gotti ha messo in evidenza, non vi è dubbio che i tempi saranno dilatati e su questo vi è un allarme del Consiglio superiore della magistratura, dei costituzionalisti

Faccio questa premessa perché la questione pregiudiziale che mi appresto ad illustrare parte naturalmente dal presupposto che il reato

messo in evidenza nella precedente lettura del Senato che risale ormai a tempo fa, questa fiducia rischia anche di mettere in discussione alcuni canoni fondamentali. Alle volte mi trovo a dire che stiamo per approvare un decreto-legge. In realtà, si tratta semplicemente di un disegno di legge che, partito dal lontano maggio del 2008 adesso sta per approdare alla sua conclusione, perché improvvisamente si è deciso di mettere la fiducia dopo che vari provvedimenti sono stati inseriti nell'ambito dello stesso.

alcune norme che in apparenza sembrano venire incontro ad esigenze di non discriminazione e di eguaglianza, finiscono con l'aggravare la situazione. Sappiamo che l'articolo 6, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 attualmente in vigore, stabilisce senza alcuna incertezza che, fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo e per quelli inerenti agli atti di stato civile o all'accesso a pubblici servizi, i cittadini stranieri devono esibire carta o permesso di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni ed iscrizioni ed altri provvedimenti di loro interesse. L'articolo 1, comma 22, lettera *g)* del disegno di legge che stiamo esaminando, modificando l'articolo 6, comma 2, del Testo unico dell'immigrazione, stabilisce l'obbligo per il cittadino straniero di esibire la carta o il permesso di soggiorno anche per i provvedimenti inerenti agli atti dello stato civile o all'accesso a pubblici servizi, prevedendo l'eccezione solo nei casi inerenti all'accesso alle prestazioni sanitarie, di cui all'articolo 35 del Testo unico sull'immigrazione, o per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Tutto questo sembrerebbe aver migliorato la situazione, ma non è così. Infatti, il comma 5 dell'articolo 35 del Testo unico sull'immigrazione, soppresso poi nel corso dell'esame al Senato in prima lettura e ripristinato, invece, alla Camera dei deputati, prevede, sì, che l'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme del soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo nei casi in cui sia obbligatorio il referto ed a parità di condizioni con il cittadino italiano. Ma questa norma deve fare i conti con il reato di illegale ingresso ed illegale soggiorno nel territorio dello Stato, perché l'applicazione delle disposizioni in esame, introdotte dalla Camera, si combina con gli effetti dell'introduzione nell'ordinamento di questo reato ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato introdotto con l'articolo 1, comma 16, del disegno di legge che modifica l'articolo 10 del Testo unico dell'immigrazione.

soprattutto in una disparità di trattamento in tema di accesso a servizi pubblici essenziali relativi a beni fondamentali tutelati dalla Costituzione da parte degli immigrati che non hanno o non hanno più un valido titolo di soggiorno. Tutto questo perché i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di denunziare, se ne vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni, un reato procedibile d'ufficio, quale è appunto quello di ingresso e soggiorno illegale (pur essendo contravvenzionale, è procedibile d'ufficio). Tutto ciò in stridente contraddizione con la norma di esenzione dall'obbligo di denunzia dello straniero irregolare da parte del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio previsto dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35.

tale obbligo i funzionari e i dirigenti delle amministrazioni delle ASL, che sono già oggi tenuti, a fini di rendicontazione, a trasmettere al Ministero dell'interno il dato sulle prestazioni erogate a stranieri in condizioni di soggiorno. Da ciò nasce chiaramente una violazione da parte della nuova normativa, pur nella modifica approvata dalla Camera, degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, proprio sotto il profilo della violazione di diritti fondamentali, di condizioni di uguaglianza, del principio di ragionevolezza e del diritto alla salute. Basta presentarsi e, in pratica, vi è l'obbligo di denunzia. Allo stesso modo, e cerco di chiudere questo discorso, ci troviamo a ragionare quando vi sono altri diritti costituzionalmente garantiti che vengono limitati; la preclusione all'immigrato irregolare del perfezionamento degli atti di stato civile, quali la registrazione della nascita, della morte, il riconoscimento del figlio naturale, il matrimonio, il diritto all'istruzione. Perché subordinare al possesso di documenti regolari, soprattutto in materia di accesso ad alcuni servizi di stato civile, già rappresenta una violazione degli articoli 2, 3, 29, 30 e 31 della Costituzione; se a questo aggiungiamo che un ufficiale di stato civile ha

La stessa identica cosa avviene per quanto riguarda il diritto all'istruzione, che gli articoli 2, 3, 30 e 34 della Costituzione riconoscono, perché anche in questo caso il figlio minore di genitori irregolari

peggiorativo e spingere ancor di più a situazioni di irregolarità. In considerazione di tali aspetti di palese violazione della Costituzione chiedo pertanto, Presidente, che non si proceda, a norma dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, all'esame del disegno di legge n. Senatrice Della Monica, non entro certo nel merito del suo intervento, come di altri, perché non è compito di chi presiede. Vorrei però fare una precisazione in merito ad un aspetto. I turni della Presidenza vengono determinati a rotazione non in relazione agli argomenti in discussione. Ritengo che questo criterio sia giusto e vada mantenuto, perché è l'unico che garantisce che ci sia uno sforzo di ruolo istituzionale della Presidenza. Inoltre, ricordo a tutti i colleghi, anche se non

parlerò soltanto di una delle questioni di illegittimità costituzionale del disegno di legge

quando stava per entrare in vigore il nuovo codice di procedura penale. Bisognerebbe chiedersi per quale ragione questo reato è stato abolito. che con il nuovo codice di procedura penale la prova veniva raccolta in dibattimento e non più durante la fase istruttoria; quindi, si sapeva perfettamente che il sistema sarebbe stato

Peraltro, questi tempi incidono anche sulla sicurezza dei cittadini e, quindi, la prima cosa che ci meraviglia quando viene reintrodotto un reato e quando ne vengono stabiliti altri è che si aggrava proprio tale situazione. della giustizia penale, e poi la sicurezza dei cittadini viene danneggiata: quanto più durano i processi tanto meno efficace è la repressione Lo sappiamo tutti: tutti chiediamo l'immediatezza e l'esecutività della pena; tuttavia ci guardiamo bene dal comportarci in modo tale che i nostri processi penali vengano definiti in tempi accettabili.

se prima del giudizio l'imputato abbia riparato interamente il danno. Badate bene, questa è una circostanza che riguarda

il perdono giudiziale e, quando poi sono trascorsi i tempi necessari, l'estinzione per effetto della sospensione condizionale della pena. Come vedete, si tratta di cause di estinzione che riguardano la generalità dei reati,

situazione di disparità assoluta, che contrasta con l'articolo 3 della nostra Costituzione, il quale stabilisce che siamo tutti uguali davanti alla legge senza distinzioni,

e togliersi addirittura lo sfizio di farlo positivamente; chi invece è povero e disgraziato dovrà subire le conseguenze di un reato punito fino a tre anni di reclusione.

ovvero quella della prestazione sanitaria che vede coinvolti cittadini stranieri. Essa è stata, per la verità, solo apparentemente risolta nelle modifiche che hanno seguito l'esame del testo, ma presenta nel combinato disposto dell'articolo 10-*bis*, laddove si prevede il reato contravvenzionale di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato dello straniero,

di segnalazione alle autorità, profili di problematicità e di incostituzionalità, laddove non si dichiara esplicitamente l'esenzione dell'obbligo di denuncia per il pubblico ufficiale o per l'incaricato di servizio pubblico dentro il servizio sanitario. Vorrei ricordare il diritto fondamentale previsto all'articolo 32 della Costituzione - la tutela della salute - e la consolidata giurisprudenza relativa, la quale afferma che va impedito in ogni modo il sorgere di situazioni prive di garanzie e di tutela, che possono in qualche modo pregiudicare l'attuazione di quel diritto. Si deve quindi evitare in modo esplicito e non soggetto a interpretazioni - per questo abbiamo posto la questione pregiudiziale - che gli obblighi di denuncia in capo a pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, connessi all'introduzione del reato di immigrazione clandestina, possano vanificare la manleva posta in capo a quegli stessi soggetti quando erogano una prestazione sanitaria.

nel presente disegno di legge, se parliamo di interventi che mirano ad accertare nuove fattispecie di reato e ad incrementare le pene per comportamenti odiosi alla comunità, per dare in buona sostanza risposta alla ragionevole richiesta di maggior severità e rigore, vi sono di certo elementi condivisibili. Penso ai reati che attengono alle fattispecie cosiddette di minorata difesa nei reati di truffa, previsti al comma 28 dell'articolo 3, alle sanzioni relative alla mutilazione genitale femminile, al comma 59 dello stesso

perché non deve derivare da questo dibattito l'idea, che va rigettata con forza, di un nostro disinteresse o di una nostra trascuratezza rispetto alle richieste di maggior sicurezza o di maggior rigore che vengono da più parti. Cos'è che, nella lettura complessiva della vicenda sicurezza, se guardiamo a questa produzione normativa, per noi non può essere considerato convincente? Innanzitutto appare una linea politica, che si traduce peraltro in norme, che, dove si pronuncia sicurezza, si legge in verità immigrazione, con la volontà di dare a quest'ultima non una risposta in termini complessivi e di regolamentazione, bensì l'immagine che l'immigrazione in fondo è come una malattia che se cureremo con determinazione prima o poi verrà debellata e scomparirà e finalmente il nostro corpo nazionale tornerà ad essere integro ed omogeneo. Allora è meglio non unire ma dividere, non integrare ma disgregare,

come si può pensare che i problemi in campo possano essere in qualche misura risolti? Si risolvono complicando chi deve chiedere un permesso di soggiorno? Si risolvono complicando l'educazione dei figli o l'accesso alle strutture sanitarie? rispondere positivamente a questa linea complessiva che si determina in questo anno di lavoro perché di fatto ci troviamo di fronte alla messa in atto di una sorta di legge speciale parallela, un sistema duale, persino a volte un diritto penale straordinario destinato agli stranieri. al di là delle singole norme che abbiamo contestato, ci appare nel suo complesso contro il dettato costituzionale, che va in un'altra direzione, che segue altre che segue altre indicazioni, che sono quelle di un progresso certamente ordinato ma che in qualche misura tenga conto della necessità di cambiamenti che possono favorire e risolvere le questioni all'interno di una società con delle politiche appropriate e mirate a risolvere i problemi stessi. Per questo e per gli altri motivi che abbiamo richiamato, chiediamo che non si passi all'esame del disegno di legge

abrogato dal Senato in prima lettura, è stato ripristinato nel corso dell'esame da parte della Camera dei deputati. È stato ricordato già dalla collega Della Monica e dal collega Galperti il fatto che si tratta di quell'articolo che vieta al personale sanitario di denunciare chi si presenta sprovvisto di permesso di soggiorno per delle cure. Come tutti sapete, questo è stato uno dei punti sui quali si è incentrato nei mesi scorsi il dibattito pubblico sul provvedimento che stiamo discutendo. Sapete che dal mondo della salute, dal mondo della sanità nelle sue diverse articolazioni professionali e associative è venuto su questo punto del disegno di legge un pronunciamento molto forte. Nel mondo del volontariato credo che non ci sia un'associazione, di quelle che si conoscono e che danno attività, che non abbia preso posizione su questo aspetto del provvedimento. Anche dalla Chiesa cattolica e da altre confessioni religiose è venuta al riguardo una posizione

che politica, che ha fatto considerare addirittura a molte persone e a tanti operatori sanitari la strada dell'obiezione di coscienza, con l'impegno a sottoscrivere dichiarazioni nelle quali affermavano di non essere disposti a dare applicazione alla nuova normativa che la maggioranza proponeva, assumendosi quindi responsabilità, prendendo una posizione ed essendo disposti a pagare prezzi seri. Perché questo è avvenuto?

La conseguenza più grave di ciò è certamente quella che colpisce le persone che non ricorreranno alle cure delle quali avrebbero avuto bisogno, venendo così private di un diritto fondamentale.

lontani dalle strutture sanitarie significa anche tenere lontana la malattia. E non credo sia necessaria una particolare specializzazione in epidemiologia per capire che questo rappresenta un problema per l'igiene pubblica, soprattutto quand'è serio il rischio che con i flussi migratori si spostino anche nuove malattie e si riduca in questo modo la possibilità di conoscerle e controllarle. Insomma, per gli operatori sanitari si sarebbe determinata una ferita profonda,

Il dibattito alla Camera ha dovuto tener conto di una protesta così ampia e del fatto che l'opinione pubblica aveva dimostrato di non condividere questa scelta, il comma 5 dell'articolo 5 del Testo unico sull'immigrazione è stato ripristinato. Tra parentesi, per quanto mi riguarda, ho riflettuto su questo fatto e penso mi insegna - in questa situazione politica in cui per tanto tempo noi uomini dell'opposizione e del centrosinistra ci siamo lasciati andare a rappresentare una presunta onnipotenza del Governo,

di questioni che aprivano una crisi e mettevano in difficoltà il rapporto con la società e la sua espressione. Ecco, questo è il punto: la marcia indietro che la maggioranza ha dovuto fare alla Camera - lo ribadisco - è un fatto positivo, che cancella una norma aberrante, ci consegna un testo che - com'è già stato fatto rilevare - apre la strada a contraddizioni ed incertezze interpretative, che rischiano di portare il problema al punto di partenza.

dell'articolo 361, che parla dell'omessa denuncia da parte del pubblico ufficiale, e dell'articolo 362, che parla di omessa denuncia da parte dell'incaricato di pubblico servizio, diventerà praticamente impossibile un'interpretazione univoca della norma e dell'obbligo o meno di denuncia da parte del personale sanitario. L'introduzione del reato di immigrazione clandestina e gli obblighi di denuncia che da esso discendono in capo ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio risultano in stridente contraddizione con la norma di esenzione dall'obbligo di denuncia dello straniero irregolare all'autorità giudiziaria prevista dal più volte citato comma 5 dell'articolo 35. Tale incertezza, e il timore che questo può determinare, in particolare in un contesto culturale nel quale ormai è evidente che c'è chi alimenta un clima di ostilità nei confronti degli immigrati, provocare lo stesso effetto: quello di creare una situazione di incertezza che allontana le persone, come gli immigrati irregolari, che hanno bisogno di cure dalle strutture sanitarie. In tal modo si torna a ledere quel diritto alla salute in nome del quale la Costituzione impone di impedire che si determinino situazioni prive di tutele, tali da pregiudicare l'attuazione di quel diritto fondamentale. È per questa ragione che, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, chiediamo di non procedere alla discussione del disegno

dell'umanità di cui dobbiamo parlare. L'umanità, sia di chi ha cittadinanza italiana, sia di chi non ce l'ha. Appassionati, senatore Saltamartini, anche della nostra Costituzione. Appassionati di questo Parlamento. Non posso credere, perché vi conosco da tanto tempo, amico Giacomo Caliendo - oso chiamarlo così - e senatore Filippo Saltamartini, che alcune delle osservazioni che abbiamo fatto non abbiano fatto breccia nella vostra razionalità. Siamo di fronte ad un testo che è stato modificato in parte dalla Camera che lo ha reso, sotto alcuni punti di vista, più controverso, ma - apro una parentesi - meno male che ci sono due Camere, perché qualche volta la resipiscenza fa bene.

Poco fa abbiamo sentito citare i medici, i dirigenti sanitari: tutte persone che a causa di una modifica che ci ha allargato il cuore quando l'abbiamo letta in realtà non provoca effetti positivi.

gli incaricati di pubblici servizi sanno di poter non obbedire alle leggi. È una bella storia in termini pedagogici! Per fare una normativa che dovrebbe rendere il Paese sicuro, perché tutti rispettano le regole,

che fosse chiarito questo elemento, perché si ha a che fare con uno dei diritti più inviolabili dei bambini - non so perché poi sottoscriviamo le Convenzioni dell'ONU - cioè l'accesso all'istruzione. L'alfabetizzazione è uno degli strumenti più elevati per riconoscere la dignità delle persone, a maggior ragione di quelle che hanno per forza bisogno della tutela degli adulti, talché quando non c'è l'adulto è lo Stato a tutelare il minore. In questo caso, i minori vengono abbandonati, perché se non possono stare a scuola dove stanno? stanno? Sono bambini che cominciano ad essere invisibili quando non possiamo denunciarli all'anagrafe e che continuano ad essere invisibili, tranne diventare accattoni, essere coinvolti nella prostituzione,

- non stiamo perdendo tempo e non facciamo perdere tempo. Crediamo che stiamo parlando di uno dei diritti più importanti. La nostra Carta costituzionale prevede il diritto allo studio perché è il diritto che qualifica la persona, che rende civili. Anche Anche tutti i dibattiti che stiamo facendo sui provvedimenti del ministro Gelmini sono intorno a questo fatto: quando la norma viene riconosciuta come strumento di promozione della persona rende le persone migliori. Quindi, attraverso la scuola noi avremo dei processi di integrazione migliori. Altro che imparare la lingua. Imparerebbero le nostre regole! A scuola si studia anche la Costituzione ed è prevista l'educazione alla cittadinanza. lasciar fuori da tutte queste opportunità, che qualificano, rispettano, riconoscono e promuovono la dignità della persona, proprio i bambini, che ne avrebbero più bisogno?

che non devono dire bugie, che non devono imbrogliare le carte e che dimostrino loro per primi che sanno rispettare le regole. Per tutti questi motivi, e molti altri sui quali potrei anch'io indugiare per raccontare, ma che i colleghi hanno già ben indicato,

ronde, particolarmente scabroso perché ci ricordiamo in molti la definizione che dello Stato moderno ha dato Max Weber: abbiamo lo Stato moderno quando abbiamo il monopolio dell'uso legittimo della forza. Quindi, non ci sono delle milizie private che spadroneggiano sul territorio, magari corrispondendo a fazioni e partiti. Il tema è stato affrontato a proposito del Libano, dopo opera la milizia di Hezbollah, una milizia di partito, che dà l'idea dei rischi cui andiamo incontro.

Nobilitare tutto ciò in nome del principio di sussidiarietà, riconosciuto dall'articolo 118, come innovato con la riforma del Titolo V, che serve ad una migliore gestione dei servizi collettivi, a cominciare dai servizi sociali, di cui nessuno nega l'utilità, tanto è vero che lo abbiamo concordemente inserito nella Costituzione,

episodi di violenza, di mancato controllo del territorio, ma per cooperare con le legittime forze dell'ordine, provocando probabilmente a tali forze più problemi nel controllare loro che non già la criminalità. Come possiamo dimenticare, per esempio, l'articolo 18, comma 2, della Costituzione che recita: «Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare»? Queste norme della nostra Costituzione sono nate per ribadire il principio fondamentale del monopolio dell'uso legittimo della forza e, non a caso, l'articolo 117, nel descrivere puntualmente le competenze di Stato e Regioni, ha solennemente stabilito che ordine pubblico e sicurezza sono materia esclusiva dello Stato. Sappiamo bene che certe cose non funzionano, che c'è uno scoordinamento tra varie forze di polizia, che abbiamo un problema di bilancio (fra l'altro, aggravato dal nostro Governo), però, l'idea di risolvere questo esternalizzando verso poteri privati di incerta definizione al confine tra le milizie e con un ruolo partitico aggrava il problema e non lo risolve. Rispetto a queste nostre preoccupazioni, l'inserimento presso la Camera dei deputati del rinvio ad un decreto del Ministero dell'interno che dovrebbe disciplinare questa norma è stato presentato come una sorta di panacea. cioè detto: avete delle preoccupazioni, è vero che ci sono forze un po' confuse o anche pericolose che si muovono sul territorio, ma vedrete che poi quando si passerà ad una fonte secondaria, quindi ad una fonte che deroga a principi costituzionali come quello dell'ordine e della sicurezza come materia esclusiva dello Stato dove c'è un'evidente riserva di legge, quando arriverà questa disciplina secondaria, essa risolverà i problemi perché sarà restrittiva quegli spazi per iniziative di persone o di gruppi non sensate verranno frenate. Ma è possibile varare una legge così delicata dicendo che i problemi ci sono, ma verranno poi risolti da una norma secondaria a seconda di come un decreto del Ministero dell'interno potrà confezionare poi la pratica attuazione della norma? La riserva di legge sancita solennemente nell'articolo 13 rispetto alla libertà personale del cittadino, che potrebbe essere intaccata da atti coercitivi di questi gruppi, viene violata così palesemente dicendo che saremmo rassicurati da una fonte secondaria. secondaria. Penso si possa fare tutto per aiutare i cittadini singoli ed associati a collaborare con le forze dell'ordine per segnalare le difficoltà, che esistono, di effettivo controllo del territorio, ma così facendo rendiamo il controllo del territorio ancora più incerto e, soprattutto, andiamo ad impattare con gli articoli 13 e 18 della Costituzione.

Il comma 23 dell'articolo 1 prevede l'applicazione delle disposizioni relative al prolungamento della durata della permanenza nei centri di identificazione ed espulsione a 180 giorni i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, anche se già trattenuti nei centri di identificazione ed espulsione alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, stabilendo quindi l'efficacia retroattiva della disposizione stessa. Questa disposizione, quindi, rappresenta un elemento di grave preoccupazione: essendo il trattenimento in un CIE una restrizione della libertà personale, ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione, a maggior ragione dovrebbe valere un principio di irretroattività per misure sanzionatorie di cui l'interessato non era a conoscenza nel momento in cui ha posto in essere il comportamento. Se è vero che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, e ciò in base all'articolo 25 della Costituzione, per rispettare il dettato costituzionale, il legislatore non può prevedere una restrizione della libertà personale con una legge che entra in vigore successivamente all'inizio del trattenimento dell'interessato. L'ingiusto e illegittimo prolungamento del trattenimento di persone già ristrette in strutture chiuse provocherà un pericoloso innalzamento del livello di tensione delle persone, con inevitabili drammatiche conseguenze. Per questo motivo, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento del Senato, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n. 733-B. *(Applausi

ma prima di entrare nel merito, poiché ritengo che questo sia un elemento che pregiudichi la costituzionalità del provvedimento, vorrei soffermarmi

estremamente gravi hanno già parlato i colleghi, in particolare per quanto riguarda il reato di immigrazione clandestina, che è un un *vulnus* gravissimo, sia per quello che riguarda la sicurezza, che in realtà questo provvedimento dovrebbe salvaguardare, sia per quello che riguarderà la vita concreta di persone in carne ed ossa, che soltanto perché immigrati diventano immediatamente fuori legge.

fuori dalla legge o anche solo fuori dalle regole della convivenza civile della comunità, ma semplicemente per il fatto di provenire da un altro Paese, di essere degli immigrati.

chi vietava di affittare case, chi diceva che i servizi pubblici non potevano più essere utilizzati, per arrivare a quella che ho ritenuto tra tutte l'ordinanza più aberrante - e mi dispiace molto che sia stato un sindaco donna a proporla - che vietava le

Probabilmente da bambini hanno frequentato la scuola dell'infanzia con i nostri figli, hanno imparato l'italiano e giocato con loro e con loro sono andati in gita scolastica alle medie.

i nomi dei ragazzi stranieri che stavano per compiere 18 anni, dicendo che voleva suggerire loro di portare i documenti, ma di fatto è stata una lista ed alcuni di questi ragazzi non sono più tornati a scuola. Possiamo pensare che questo possa servire alla sicurezza? Che questo renda più sicuro il nostro Paese? Ma non dovrebbe essere tutto il contrario, non dovremmo incentivare questi ragazzi ad andare a scuola e ad essere inseriti in percorsi formativi?

i requisiti e la sentenza della Corte costituzionale aveva chiarito che andavano considerati elementi alternativi e non concorrenti. Quindi, per questo motivo ricompreso nella filosofia che ho cercato di descrivere dall'inizio e che

norma che modifica l'articolo 6, comma 2, del Testo unico sull'immigrazione, prevedendo l'obbligo per il cittadino straniero di esibire la carta o il permesso di soggiorno anche per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all'accesso ai servizi pubblici, facendo eccezione solo nei casi inerenti l'accesso alle prestazioni sanitarie e quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie. Sull'ingiustizia, dannosità, negatività ed incostituzionalità di questa norma si sono già pronunciati molti colleghi del Gruppo del Partito Democratico e dell'opposizione. Quindi mi soffermerò nell'illustrazione della pregiudiziale non tanto sull'aspetto generale della norma, quanto sulle eccezioni che sono introdotte alla stessa, in particolare sul fatto che risulterebbero esenti da questa richiesta le prestazioni sanitarie e scolastiche obbligatorie. Innanzitutto, chiedo ai colleghi senatori se è possibile ragionare di scuola, di scuola dell'obbligo, quella che forma e che dà pari opportunità a tutti i bambini in termini di prestazioni scolastiche obbligatorie. La scuola non è un servizio a domanda individuale, non è una prestazione ma un ordinamento della Repubblica che ha il compito di condurre all'istruzione, alla crescita, all'educazione tutti i bambini, tutti ragazzi e dare loro quelle opportunità che che sono assolutamente diversificate, a seconda della famiglia di provenienza dei ragazzi stessi. Dunque, la scuola è una istituzione della nostra Repubblica e, come tale, non è

a seconda delle capacità, della cultura che ha e, quindi, sostanzialmente con un richiamo alla differenziazione nella scelta. Ciò è l'esatto contrario dell'obiettivo che la scuola deve perseguire: non favorire i già favoriti ma, al contrario, dare di più a chi ha di meno. D'altra parte, proprio don Milani ce lo ha illustrato con grande efficacia. La scuola deve essere il luogo dove viene dato di più a coloro che hanno di meno. Invece, in questa concezione, ciò non c'è nel modo più assoluto. Soffermiamoci su un fatto: prestazioni scolastiche obbligatorie. In concreto, con la legge finanziaria 2007, il Governo Prodi ha innalzato l'obbligo di istruzione a 16 anni. Vorrei pensare che questa norma faccia riferimento all'obbligo dell'istruzione e quindi ragioni sul fatto che fino a 16 anni ci si può iscrivere a scuola, senza la condizione di presentare il proprio permesso di soggiorno; dopo, invece, ciò non sarà pertanto al paradosso, all'ingiustizia e all'inspiegabilità dal punto di vista della logica del fatto che un ragazzo fino a 16 anni possa frequentare un percorso d'istruzione e,

capaci ed i meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi negli studi. In questo caso, per i ragazzi stranieri privi di permesso di soggiorno c'è invece uno sbarramento; si frequenta la scuola dell'obbligo e nulla più. Tra l'altro, vorrei che il Ministro ci dicesse qual è l'indicazione dell'obbligo, perché un provvedimento da lei stessa attivato farebbe pensare che l'obbligo alla terza media, laddove il ragazzo deve poi scegliere tra un percorso di istruzione e un percorso di istruzione e formazione professionale di carattere regionale, quindi uscire dalla scuola. Peraltro, qui non è indicato cosa accadrebbe a questo ragazzo. Voglio ancora sottolineare come

ha richiesto a tutti i ragazzi che dovevano essere ammessi all'esame di maturità, un codice fiscale validato dall'Agenzia delle entrate. delle entrate. Un codice fiscale lo si può costruire con grande facilità da parte di ognuno, ma il fatto che per essere ammessi all'esame di maturità occorra un codice fiscale validato dell'Agenzia delle entrate ha suscitato da parte di molti di noi, e soprattutto da parte di molti dirigenti scolastici, studenti, associazioni e sindacati, grande allarme, perché si è pensato che già prima dell'approvazione della legge questa venisse, nei fatti, applicata relativamente all'ammissione all'esame di maturità, poiché non veniva precisato cosa sarebbe accaduto al ragazzo che fosse stato privo del codice fiscale validato dall'Agenzia delle entrate. Siamo in un'Aula parlamentare: vorrei chiedere ad ognuno di noi che senso ha richiedere la validazione dell'Agenzia delle entrate di un codice che dovrebbe servire semplicemente per creare un'anagrafe degli studenti che partecipano e sono ammessi all'esame di maturità. Dopo una grande sollevazione, e soprattutto dopo i casi che concretamente si sono presentati e che sono stati evidenziati dalla stampa di ragazzi bravissimi che avevano frequentato tutto il liceo o che stavano ancora frequentando la scuola quando è emerso il problema, il

il principio di uguaglianza di diritto, laddove tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, ma anche dell'uguaglianza di fatto laddove si dice che la Repubblica deve promuovere tutte le condizioni che evitino il dispiegarsi, a seguito di differenze di varia natura, di condizioni di disparità.

Aggiungo, a seguito di questo mio ragionamento sulla scuola dell'obbligo, che una discriminazione gravissima si produrrebbe anche per ciò che riguarda l'iscrizione all'università, perché, non solo non si potrebbe continuare il percorso di istruzione, ma, a seguito di tale norma, anche chi avesse già i titoli per iscriversi all'università

Tra le diverse disposizione del disegno di legge che generano rilevanti perplessità sotto il profilo della legittimità costituzionale (come hanno richiamato molto puntualmente i colleghi), vorrei sottolineare l'attenzione del Senato sul comma 18 dell'articolo 1,

possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie». In questa dizione credo di poter rilevare in modo fondato due questioni che hanno a che vedere con l'obiezione di costituzionalità. La prima, comune anche al testo precedente, riguarda l'indeterminatezza della norma dal punto di vista del riferimento. Alludo non viene specificato cosa si intenda per condizioni igienico-sanitarie dell'immobile a scopo abitativo. Ad esempio, non si cita il Testo unico in materia di edilizia

cioè quella condizione di cui è privo il 50 per cento del patrimonio immobiliare italiano, compreso forse il palazzo da cui stiamo decidendo queste restrizioni.

quale però ha a che vedere con i diritti di cittadinanza garantiti su tutto il territorio nazionale: un cittadino, ovunque risieda, ha il diritto di chiedere la residenza e i requisiti normalmente richiesti hanno a che vedere con i suoi requisiti soggettivi.

è stata eliminata e apparentemente ammorbidita. Il problema è che, a proposito di una questione che ha a che vedere con i diritti di cittadinanza (perché attraverso la residenza si acquisisce, ad esempio, l'accesso all'anagrafe e la possibilità di richiedere una carta d'identità, ossia di essere considerati, ancorché provvisori, cittadini di quel comune),

Intanto non si chiarisce quando e a quali condizioni scatti tale verifica e nemmeno si chiarisce cosa succederà dopo.

di volta in volta, se fare la verifica o non farla e quali criteri far valere o meno. Avrà la residenza chi vive in uno di questi deliziosi

casi non ci saranno i requisiti? Si sta creando una soggettività, che è assolutamente contraria

che tale norma abbia di mira gli stranieri. Se avessimo voluto stabilire che non vogliamo dare la residenza alla gente che vive nelle *roulotte*,

un'abitazione? L'antibagno, che non ha nessuno? Gli stranieri che vivono nelle nostre amate case di ringhiera milanesi

stato sottolineato anche per altre norme - con ipocrita coerenza l'obiettivo di rendere la vita difficile o impossibile non ai clandestini e nemmeno ai cosiddetti irregolari (categoria che sta nascendo con questa maggioranza e questo Governo, perché non sanno dove mettere 650.000 clandestini prodotti dalla cosiddetta legge Bossi‑Fini, aprendo una distinzione interessante fra clandestini ed irregolari),

Invece c'entra, perché in realtà, come hanno già detto alcuni colleghi, state approvando delle norme inutilmente crudeli, inutili rispetto all'obiettivo o, peggio, che rendono la presenza degli stranieri un elemento di maggiore insicurezza. Norme come questa, infatti, comportano il rischio di avere una massa indeterminata di precari sempre ricattabili,

attira immigrazione di bassa qualifica, che ci crea più problemi e mette queste persone, che non trovano uno Stato che sappia dir loro quali sono i loro diritti e garantirli, nelle mani di chi organizza la tratta

colleghi senatori, intendo sollevare, illustrandola, una questione pregiudiziale sulla norma di cui alla lettera *l)* del comma 22 dell'articolo 1.

almeno dal punto di vista del *drafting* legislativo. Questa norma non era nata così quando era stata licenziata per la prima volta infatti reintrodotto vecchi concetti che erano propri di alcune leggi finanziarie, in cui ad un certo punto, per far passare di tutto e di più, veniva tutto compresso, rendendo difficile la trasparenza, che dovrebbe essere uno degli elementi principali della norma.

sono propri i colleghi di maggioranza, perché quando ci troviamo nelle condizioni per cui un Governo continua ad adottare provvedimenti che non permettono mai un'interlocuzione né da parte delle delle Commissioni, né da parte di coloro che dovrebbero essere i primi ad avere un rapporto dialettico con il Governo stesso, cioè i colleghi della maggioranza, significa che si continua a stravolgere se non altro quel principio della divisione dei poteri che

faccio riferimento alla lettera *l)*, del comma 22, dell'articolo 1, che dispone l'estensione del termine massimo del trattenimento dello straniero nei centri per l'identificazione ed espulsione dagli attuali due mesi a sei mesi «in caso di mancata cooperazione al rimpatrio del cittadino del Paese terzo interessato o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi». Permettetemi subito di aprire una seconda chiosa: si tratta di una norma che era presente nel provvedimento che avevamo analizzato in questa sede (e mi ricollego al tema dell'utilizzo e abuso dello strumento della fiducia). Questa Assemblea, a scrutinio segreto, aveva bocciato tale norma. Il Governo, che doveva pagare un pegno alla Lega Nord che di questa norma aveva fatto una bandiera (perché qui non andiamo avanti cercando di fare norme di carattere generale che badano al bene pubblico, ma cerchiamo di assecondare gli di assecondare gli istinti che in una parte della maggioranza fanno sì che possano essere vendute all'esterno alcune norme che io definisco norme manifesto; ricordo che è stata bocciata dal Senato, poi è stata reintrodotta dalla Camera e anche lì è stata bocciata a scrutinio segreto),

potesse essere soddisfatta (si era in tempi pre-elettorali) rispetto ad un'aspettativa che per loro rappresentava una bandiera. Queste sono motivazioni politiche che - permettetemi - alla sola lettura di quello che deve essere il testo finale non possono non evidenziare aspetti che fanno sì che si sottolinei molto di più l'apparire, il voler dare un senso di risposta formale a problemi che non si risolvono, che vengono ingenerati nella pubblica opinione, rispetto ai quali si fa finta di dare delle risposte. Questo lo si capisce tanto più se si pensa che tale disposizione è strettamente collegata con la norma di cui al comma 16 dell'articolo 1, che punisce

ogni volta si diceva che si puniva di più, ma poi non si vedeva se c'era l'effettività della pena, sempre secondo la logica di cui ho detto prima), non fa altro che criminalizzare quelle che sono mere condizioni personali e presenta molteplici profili di illegittimità costituzionale. La norma è anzitutto priva di un fondamento giustificativo poiché la sua sfera applicativa è destinata a sovrapporsi integralmente a quella dell'espulsione quale misura amministrativa,

si è cercato di creare una specie di risposta fittizia alla domanda di sicurezza. Quest'ultima veniva ritenuta come elemento fondamentale per la proposta politica che la maggioranza aveva fatto al Paese

elementi meritevoli di una tutela di tipo penale né tanto meno giustificano l'estensione del termine massimo del trattenimento dello straniero nei centri per l'identificazione e l'espulsione dagli attuali due mesi a sei.

il sistema nel suo insieme non sta più in piedi:

Queste riflessioni portano ad accelerazioni pericolose su molti temi e ad un'identificazione della condizione del migrante come quella

cui si danno risposte di carattere propagandistico. E tutto questo lo si fa calpestando la Costituzione. Per questi motivi, ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, chiediamo di non procedere all'esame del disegno di legge n.

Presidente, ho chiesto la parola per intervenire

che interloquisca con il Governo. Infatti, per uscire dalla crisi è chiaro che sono necessari degli investimenti pubblici; ed è chiaro che la politica deve fare la sua parte,

negoziazione con la FIAT: che non venga assolutamente toccato nessuno stabilimento. Signor Presidente, in queste ore nello stabilimento di Termini Imerese ci sono delle civili, ma accorate proteste. E questo stabilimento ha delle potenzialità enormi sia in riferimento

Ieri pomeriggio a Catania, nella zona centrale, davanti a Villa Bellini, i Carabinieri sono intervenuti in forze presso lo *stand* dell'Associazione radicale «Certi Diritti» per verificare se effettivamente si manifestavano turbamenti o atti osceni, come segnalato da un cittadino. Allo *stand* della suddetta Associazione radicale, allestito per promuovere il *Gay pride* siciliano che si svolgerà sabato 4 luglio, venivano semplicemente distribuiti volantini informativi della campagna di affermazione civile in cui si chiede a

dispiegando mezzi e uomini, e hanno potuto ricevere il materiale dell'Associazione stessa, che però, a questo punto, credo chieda l'immediata verifica della regolarità delle procedure (la delegazione radicale del Gruppo del Partito Democratico presenterà un'interrogazione parlamentare in tal senso), a partire dall'identificazione di chi ha procurato l'allarme. Dico tutto ciò perché la settimana scorsa a Napoli una ragazza ventiseienne, dal nome Maria Luisa, nel tentativo di difendere un amico omosessuale aggredito da sconosciuti, dopo aver chiamato il «113», che non rispondeva, è stata portata all'ospedale per le percosse subite. In molti parlamentari abbiamo firmato un appello al Presidente della Repubblica perché le venga conferita

di chi vive la propria vita in maniera diversa per questioni di identità di genere e orientamento sessuale: cioè, qui l'omofobia è la vera emergenza e non c'è una sola misura, in tutti i provvedimenti che ci avete proposto da quindici mesi a questa parte, che tuteli questo gruppo di persone.

a come l'Italia uscirà da questa situazione di crisi. Quindi, condivido pienamente le sue preoccupazioni. La Presidenza chiederà al Ministro dello sviluppo economico di riferire in Aula. In ogni caso, come lei ha già detto, se il Gruppo del Partito Democratico presenterà una mozione specifica, la Presidenza